L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B ai Resoconti della seduta. Avverte

ha approvato il calendario dei lavori per la settimana dal 3 al 5 maggio. Rimane confermato il calendario per la settimana corrente che prevede l'esame del decreto-legge recante interventi in favore della cultura e altre disposizioni urgenti. Nella prossima settimana l'Assemblea non terrà seduta. Le Commissioni potranno convocarsi in relazione alle esigenze dei rispettivi programmi dei lavori, con particolare riferimento all'esame del Documento di economia e finanza 2011. Pertanto, l'Assemblea riprenderà i propri lavori martedì 3 maggio, alle ore 17, con all'ordine del giorno l'esame del Documento di economia e finanza 2011, per il quale si è proceduto alla ripartizione dei tempi tra i Gruppi. Le proposte di risoluzione dovranno essere presentate entro la fine della discussione generale, mentre il termine per gli emendamenti alla risoluzione accolta dal Governo sarà stabilito in relazione all'andamento dei lavori. Il calendario di tale settimana prevede inoltre il seguito delle mozioni sulla razionalizzazione della rete diplomatico-consolare italiana e sugli stabilimenti balneari. Ricordo inoltre che il Parlamento in seduta comune è convocato

Presidente, da qualche giorno è in atto uno scontro durissimo tra il Presidente della Camera e il Presidente del Consiglio, che nasce da una campagna molto violenta che il Presidente del Consiglio ha messo in atto da ormai molti mesi contro la magistratura italiana. Ed io trovo singolare, veramente singolare, che il Parlamento non si occupi di questa vicenda politico-istituzionale. Mi permetta di introdurre l'argomento. Vorrei ricordare al Senato qualcosa che ho potuto leggere questa mattina, come tutti voi, e a cui attribuisco una grandissima importanza. È la lettera del figlio del giudice Galli pubblicata oggi sul «Corriere della Sera», che inizia così: «Milano, 19 marzo 1980: Guido Galli, giudice istruttore presso il tribunale di Milano, cade assassinato dai terroristi di Prima Linea. Milano, aprile 2011: decine di manifesti recanti la scritta "Via le Br dalle Procure" fanno bella mostra per le vie cittadine. 19 marzo 1980: un bambino di 12 anni piange disperato il padre ucciso. Aprile 2011: un uomo di oltre quarant'anni è costretto a leggere manifesti infamanti contro «quelle procure» che guidarono il Paese oltre la devastazione del terrorismo. Gli attacchi che da mesi si susseguono contro i magistrati, e soprattutto contro la Procura di Milano, toccano il culmine con un'accusa verso quei giudici il cui solo torto è di far rispettare le leggi e applicare la giustizia. La delegittimazione sistematica di un'intera categoria, da parte di una classe politica la cui irresponsabilità è, forse, inferiore solo alla follia di chi stampa certi manifesti, non fa altro che indebolire le istituzioni e rendere più vulnerabili tutti noi. Quale reazione a certi messaggi da parte di chi ci governa? Nulla, o poco più: il vuoto totale. C'è amarezza in chi, tanti anni fa, ha visto il proprio padre assassinato dai terroristi e oggi, nella città in cui vive, legge certe parole. Ma c'è anche la consapevolezza che, così come allora Guido Galli cadde con il Codice in mano, oggi tanti altri magistrati, tenaci e coraggiosi, con quello stesso Codice applicano le leggi. Quel bambino oggi sa che le sue sorelle maggiori, tutti i giorni, sono lì, nel Tribunale di Milano, nella "Procura delle Br", per permettere a lui, e a tutti noi, di poter vivere in un Paese giusto, libero e democratico».

che questa lettera dovrebbe invitare il Parlamento ad occuparsi del tema che sta dilaniando il nostro ordinamento costituzionale e dividendo due cariche dello Stato di così grande rilievo per una democrazia, il Presidente della Camera dei deputati e il Presidente del Consiglio dei ministri,

recante disposizioni urgenti in favore della cultura, in materia di incroci tra settori della stampa e della televisione, di razionalizzazione dello spettro radioelettrico, di moratoria nucleare, di partecipazioni della Cassa depositi e prestiti, nonché per gli enti del Servizio sanitario nazionale della regione Abruzzo***

*relatore*. Signor Presidente, signori del Governo, onorevoli colleghi, il disegno di legge n. 2665 giunge in Assemblea dopo un dibattito costruttivo e approfondito presso le Commissioni riunite 5a e 7a, nel quale sono stati affrontati nel dettaglio tutti i temi contenuti nel testo. Per le parti di competenza della 7a Commissione il provvedimento era davvero molto atteso: da tempo infatti era stata sottoposta al Governo l'esigenza non più procrastinabile di recuperare le risorse per i beni culturali, che oggettivamente rischiavano il collasso finanziario, dopo le diminuzioni di spesa della manovra estiva dello scorso anno. La necessità e l'urgenza del decreto sono quindi anzitutto motivate proprio dagli articoli 1 e 2, per cui non si può non riconoscere lo sforzo economico compiuto dal Governo per assicurare i finanziamenti al comparto. L'articolo 1 incrementa infatti, a decorrere dal 2011, il Fondo unico per lo spettacolo (FUS) di 149 milioni all'anno, aumentando la dotazione dell'anno in corso che era pari a circa 258 milioni di euro in base all'ultima legge di stabilità e ritornando così ai livelli del 2010.

Il FUS, unica fonte di sostentamento per molti operatori, aveva infatti bisogno di nuova linfa, anche in vista dell'attuazione di importanti provvedimenti di riordino come quello sulle fondazioni lirico-sinfoniche. Del resto, la filosofia del Governo è stata quella di far precedere l'attribuzione di nuove risorse da procedimenti di riorganizzazione, nell'ottica di incentivare le gestioni efficienti, di ristabilire le condizioni di funzionalità e favorire, nel contempo, un'adeguata razionalizzazione della spesa, ivi compresa la stipula di un nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro proprio per gli enti lirici. L'articolo 1 incrementa altresì per 80 milioni di euro la dotazione del Ministero per la manutenzione e la conservazione dei beni culturali e di 7 milioni di euro il finanziamento destinato agli enti vigilati dal Dicastero stesso, quali la Biennale di Venezia, la Triennale di Milano, la Quadriennale di Roma, il Festival dei Due Mondi di Spoleto, Italia Nostra, il Fondo ambiente italiano-FAI, e altri Una conquista senz'altro rilevante è la messa a regime degli incrementi di risorse, che pertanto non si configurano come interventi *una tantum* ma danno certezze al comparto; a conferma di ciò, l'articolo 1, comma 2, esclude il FUS e le risorse per i beni culturali dai tagli lineari che potranno essere operati nel caso in cui gli introiti della vendita delle radiofrequenze fossero inferiori alle aspettative. Durante l'esame nelle Commissioni sono stati presentati circa 90 emendamenti agli articoli 1 e 2 (di cui tuttavia circa un terzo inammissibili) che riguardano più strettamente la 7a Commissione del Senato: indubbiamente si è registrata un'attenzione notevole di tutti i parlamentari, soprattutto in vista di un mutamento della copertura, per ciò che concerne l'articolo 1, e di una specificazione degli interventi per Pompei in ordine all'articolo 2. Il fatto che fino ad ora non siano state apportate modifiche al testo non comporta che non siano allo studio del Governo - e io me lo auguro - soluzioni eventualmente migliorative del testo: mi riferisco in particolare al tema della copertura delle risorse per i beni culturali, che grava sull'accisa della benzina. Nella discussione le proposte sono state molteplici, imperniate tanto sulla ricerca di diversi ambiti di innalzamento della pressione fiscale quanto sulla riduzione delle spese, ma non è stato possibile valutarle più attentamente anche a causa dell'assenza del parere della Commissione bilancio sugli emendamenti, che avrebbe senz'altro verificato la fattibilità di ciascuna opzione e dunque aiutato i relatori nell'espressione dei pareri. Mi rimetto dunque alle decisioni dell'Esecutivo, rilevando però che la copertura attuale garantisce la stabilità delle risorse, che rappresenta - come si è detto - un punto irrinunciabile. In altri casi, le modifiche al provvedimento miravano a destinare una parte delle risorse ad alcuni soggetti o eventi specifici, come ad esempio il Museo della scienza e della tecnologia di Milano, il Festival di Verdi o le celebrazioni relative alla conclusione della Grande guerra. Per queste fattispecie, che configurano una rimodulazione dei fondi complessivamente recuperati dall'Esecutivo in favore dei beni culturali, mi rimetto al Governo affinché ne valuti il possibile accoglimento. Segnalo peraltro che altre proposte, pur essendo anch'esse in larga misura afferenti al macrosettore dei beni culturali, non sono state - a mio avviso opportunamente - ritenute ammissibili dalla Presidenza, dato che risultavano comunque estranee all'oggetto proprio del decreto-legge. Mi riferisco ad esempio agli emendamenti che, modificando il decreto-legge n. 78 del 2010 (la cosiddetta manovra economica della scorsa estate), agevolavano a vario titolo gli enti culturali, sottraendoli dagli obblighi di riduzione delle spese. Si è cercato dunque di mantenere una linea direttrice univoca, in modo da focalizzare l'attenzione su un tema specifico evitando di introdurre surrettiziamente misure di carattere ordinamentale. Quanto agli emendamenti all'articolo 2, molti dei quali finalizzati a circoscrivere l'attività della società ALES spa, desidero ricordare che essa costituisce uno strumento operativo del Ministero per i beni e le attività culturali, pienamente rientrante nella fattispecie delle società *in house*, anche in virtù dell'articolo 26 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che ha trasferito al Dicastero l'intera partecipazione azionaria della società stessa. Del resto, risulta in corso un processo di razionalizzazione della struttura affinché l'attività da essa posta in essere non sia esclusivamente finalizzata all'assistenza sociale ai lavoratori socialmente utili, ma possa concorrere alla risoluzione delle urgenti problematiche che affliggono l'area archeologica di Pompei. L'obiettivo del decreto-legge in questo campo resta quello di accelerare le misure in favore di un'area particolarmente meritevole di tutela, nel quadro dei principi costituzionali. Relativamente ad altre proposte, come ad esempio quelle che dispongono la separazione della Soprintendenza speciale tra quella archeologica di Pompei e quella museale di Napoli, reputo che il carattere ordinamentale ne impedisca un'introduzione in questa sede, ma auspico che siano attentamente valutate in un successivo provvedimento.

il decreto-legge in esame si compone - come è già stato evidenziato - di sette articoli, ognuno dei quali contiene norme indipendenti tra loro, che rispondono ad esigenze emerse nel dibattito parlamentare sviluppatosi negli ultimi mesi a partire dalla legge di stabilità, esigenze condivise e portate avanti da larga ed autorevole parte dell'opinione pubblica ed anche da importanti esponenti delle istituzioni del Paese. Nell'esame in Commissione si è tenuto fermo il principio di non uscire dalle materie contenute nei singoli articoli, principio declinato nel giudizio di ammissibilità dato dai presidenti Possa e Azzollini (che voglio ringraziare per il prezioso lavoro svolto), ma anche nel lavoro di esame degli emendamenti in Commissione che, anche a causa di tale rigida preposizione, sono stati tutti respinti. Io credo che tale principio sia da tenere fermo anche nel lavoro che iniziamo oggi in Aula, al fine di non stravolgere le norme molto puntuali del decreto, memori di quello che è accaduto con il precedente decreto "proroga termini", signor Presidente, dove il Parlamento è stato messo sotto accusa per la sua eccessiva attività emendativa. Detto questo, da parte dei relatori, della maggioranza, ma credo anche del Governo, c'è la disponibilità a valutare quelle proposte che possano portare un serio contributo e miglioramento al testo in esame. Sul merito dei primi due articoli ha già relazionato il collega Asciutti, ma visto che il dibattito in Commissione si è soffermato molto sulla copertura dei 236 milioni di euro di incremento del Fondo unico per lo spettacolo e ci sono state proposte di copertura alternative, voglio brevemente sottolineare che la scelta di aumentare l'accisa sui carburanti è certo dolorosa e discutibile dal punto di vista della politica di bilancio e dell'impatto sull'economia, ma rappresenta una scelta seria che dà certezza al Paese di una copertura pluriennale ad una misura chiesta da tutta l'opinione pubblica, come anche i lavori di Commissione hanno evidenziato. Con l'articolo 3 si provvede alla proroga al 31 dicembre 2012 del divieto, previsto dal testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, per i soggetti che esercitano l'attività televisiva in ambito nazionale attraverso più di una rete, di acquisire partecipazioni in imprese editrici di giornali quotidiani o partecipare alla costituzione di nuove imprese editrici di giornali quotidiani, esigenza tra l'altro evidenziata in una recente segnalazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Si è voluto in tal modo adeguare la normativa all'evoluzione tecnologica digitale terrestre, satellitare e via cavo, rendendo più efficace la tutela della concorrenzialità e del pluralismo dei mezzi di informazione, garantendone, da una parte, la diversificazione e consentendo, dall'altra, la partecipazione al mercato di settore di più imprese di comunicazione, facenti capo a una pluralità di soggetti, anche alla luce del confronto con i principali Paesi europei.

per il passaggio al digitale terrestre al 30 settembre 2011, nonché la contestuale anticipazione del termine della assegnazione dei diritti di uso definitivi relativi alle frequenze radiotelevisive al 30 giugno 2012. In aggiunta, si prevede che, per quanto concerne le frequenze radiotelevisive in ambito locale, il Ministero dello sviluppo economico predisponga, per ciascuna area tecnica o regione, una graduatoria dei soggetti legittimamente abilitati alla trasmissione radiotelevisiva in ambito locale che ne facciano richiesta, sulla base di criteri obiettivi, quali Si tratta di un passaggio delicatissimo

È bene sottolineare che nel corso dei lavori in Commissione, su opportuna richiesta dell'opposizione, il Governo ha fornito l'entità degli accantonamenti per ogni Ministero e si è riservato di fornire un ulteriore approfondimento (arrivato

L'articolo 5 provvede alla sospensione per un anno dell'efficacia di alcune disposizioni del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, con particolare riguardo alle procedura per la localizzazione e la realizzazione nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare. La moratoria di un anno sul nucleare viene decisa al fine di acquisire ulteriori evidenze scientifiche sui parametri di sicurezza, anche in ambito comunitario, in relazione alla localizzazione, realizzazione ed esercizio sul territorio nazionale di impianti di produzione di energia nucleare. La moratoria non riguarda le procedure per la localizzazione, la costruzione e l'esercizio del deposito nazionale destinato allo smaltimento a titolo definitivo dei rifiuti radioattivi, del parco tecnologico e delle relative misure compensative. Con l'articolo 6, per le sole aziende sanitarie locali della Regione Abruzzo, si provvede alla modifica del parametro annuale su cui computare il limite percentuale della spesa sostenuta per il personale con contratti a tempo determinato o di collaborazione coordinata e continuativa, degli eventi sismici occorsi nel mese di aprile 2009. In tale contesto, anche in coerenza con il programma operativo per il rientro del disavanzo sanitario della Regione Abruzzo, si demanda l'effettiva disciplina della fattispecie alla fonte dell'ordinanza di protezione civile, i cui eventuali oneri potranno essere coperti

volto ad ampliare l'oggetto sociale della Cassa depositi e prestiti spa oltre l'attività di finanziamento tipica della società, come delineata dal comma 7 dell'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, per comprendere l'assunzione di partecipazioni in società la cui attività è considerata strategica per gli interessi nazionali, o per il settore in cui operano, o per la dimensione della società o, infine, per la rilevanza della filiera.

Viene previsto che l'acquisizione delle partecipazioni può avvenire in via diretta, o attraverso società veicolo o fondi di investimento, dei quali Cassa depositi e prestiti spa abbia sottoscritto quote, e che il *funding* potrà avvenire anche tramite le risorse del risparmio postale. Della riforma della Cassa depositi e prestiti si parla da tempo, ma ora più che mai è opportuno attuarla, allo scopo di rafforzare le strutture di un sistema che necessita di incentivi e correttivi per ricominciare a crescere. La Cassa depositi e prestiti è storicamente un'istituzione che persegue il fine di finanziare lo sviluppo della nostra economia, impiegando risorse a sostegno del settore produttivo e delle opere strategiche del Paese, contribuendo tra l'altro alla stabilità finanziaria e alla crescita europea, in un'azione condivisa con gli altri investitori dell'Unione aventi le medesime finalità istituzionali. Ecco perché è stato necessario ampliare il suo mandato, aggiungendo alla sua originaria funzione di cassa di riserva statale e istituto di finanziamento degli enti locali un respiro più ampio, allargando i suoi orizzonti istituzionali, aprendo linee di credito a lungo termine per la realizzazione di grandi progetti infrastrutturali, per la ricerca, per le nuove tecnologie (in sintesi, per mettere il Paese in condizione di dare una risposta adeguata alle sfide e alle necessità imposte dalla ripresa e da un'economia globalizzata) e aggiungendo ai noti compiti storici la partecipazione della Cassa depositi e prestiti nelle aziende nazionali di interesse strategico: certo, a condizione, come indicato nel parere nel parere della Commissione bilancio, che siano aziende sane, perché non si vuole andare in soccorso a traballanti e difettosi carrozzoni, né ricreare uno "Stato padrone", come paventato da alcuni detrattori della riforma. La *ratio* dell'intervento di trasformazione è piuttosto la creazione di un meccanismo alternativo per il credito agli investimenti, a sostegno delle attività produttive e del *made* *in Italy*, per diventare più grandi e competere ad armi pari con i concorrenti stranieri. Il modello è quello francese, ed anche quello tedesco, entrambi perni di efficienti circuiti di sviluppo economico. La creazione di un Fondo che faciliterà senza dubbio l'accesso alle risorse finanziarie, consentendo alle imprese di investire su qualità e sostenibilità, rendendone più dinamiche le strutture finanziarie e più lungimiranti i piani e i progetti, potrà funzionare se si perseguiranno reali finalità produttive estranee ai processi di degenerazione e di scontro della politica. Nel dibattito in Commissione sono emerse varie proposte dell'opposizione, si è insistito sui rischi di una simile trasformazione di Cassa depositi e prestiti ed è per mitigare tali rischi che si è deciso di aprire, cioè in Aula, a proposte emendative che aumentino, ad esempio, il controllo delle Commissioni parlamentari su questo passaggio fondamentale

su cui in questa sede si può ragionare, è quello che metterebbe in norma una precisa partecipazione della Cassa depositi e prestiti alle imprese che si occupano di gestione di reti di energia e di infrastrutture,

e forse addirittura serve a coprire altre misure che noi critichiamo, come risulterà dalla discussione che seguirà. È il difetto dei cosiddetti decreti *omnibus*. abbiamo salutato la decisione di destinare risorse a settori della cultura come una vittoria di quei mondi che, per mesi, hanno denunciato abbandono e incuria da parte del Governo. Mai si era vista una protesta così diffusa e coinvolgente, rappresentata da figure indiscusse e prestigiose in tutti i settori. In quei giorni l'unico interlocutore capace di ascoltare è stato il presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano. Dal Governo sono venuti solo silenzi o battute ironiche. Le nostre istituzioni più preziose sono state lasciate in una lenta agonia, dal cinema al teatro, alla musica, alla lirica, per non parlare degli enti culturali, di archivi e biblioteche pubbliche e private. Le risorse che ora vengono stanziate sono, dunque, tanto necessarie ad assicurare un futuro alle istituzioni culturali, quanto insufficienti. Qualcuno ha spiegato la svolta del Governo come una delle condizioni per poter realizzare l'avvicendamento che era stato concordato proprio al Ministero per i beni e le attività culturali. Quali che ne siano state le ragioni, è chiaro a tutti che si è trattato di una marcia indietro rispetto ad atti precedenti e ai tagli insostenibili di cui la cultura è stata oggetto in tutto l'arco di governo del centro destra. scelte di corto respiro, che rientrano in una visione della politica economica del Ministro del tesoro e dell'intero Governo, che non investe sullo sviluppo, ma si limita a contenere la spesa e a tagliare risorse anche in settori cruciali come la formazione, la ricerca, l'innovazione: il sapere e la cultura, appunto. Si pensa di poter abbandonare interi settori culturali al mercato, di affidarli al privato. Ma la storia e l'esperienza dimostrano che così non può essere: per svilupparsi, la cultura ha bisogno prioritariamente dell'investimento pubblico. Un recente rapporto di Federculture documenta come gli investimenti privati si riducano se si riducono quelli statali. Infatti, in concomitanza con i tagli alle risorse pubbliche, nel 2009 i privati hanno investito il 30 per cento in meno rispetto al 2008 e le fondazioni bancarie hanno erogato per la cultura il 20,5 per cento Ora le risorse vengono parzialmente reintegrate rispetto al 2010, quando già avevano subito tagli rispetto all'anno precedente. I dati di partenza avevano già un segno meno. Per il Fondo unico per lo spettacolo, lo stanziamento previsto nel disegno di legge dì stabilità per l'anno 2011 era pari a soli 258,6 milioni di euro, vale a dire il 36 per cento in meno rispetto al dato assestato del 2010, che era pari a 416,6 milioni di euro. Dunque, era stato toccato il minimo storico, che avrebbe portato a morte sicura istituzioni che fanno la storia e l'identità del nostro Paese, cinema, il teatro, la musica, la danza, le fondazioni lirico-musicali, con conseguenze drammatiche anche sul piano dell'occupazione e dell'impoverimento dell'economia che si fonda sull'indotto. Se si osserva il grafico relativo agli stanziamenti per il Fondo unico per lo spettacolo nel corso degli anni, si nota facilmente che essi toccano le punte più elevate durante i Governi di centrosinistra e quelle minime durante i Governi di centrodestra. E semplicemente un fatto. È un fatto che, durante i Governi di centrodestra, le voci del bilancio che riguardano cultura, cinema, spettacolo sono sempre con il segno meno. Ma mai si erano toccate punte così basse come quest'anno. Quanto agli 80 milioni stanziati per i Beni culturali, costituiscono anch'essi un reintegro minimo di tagli che si sono sommati nelle varie manovre economiche del triennio. Ve li ricordo. Nel disegno di legge di stabilità per l'anno 2011, rispetto alle previsioni assestate per l'esercizio finanziario 2010, lo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali presenta una riduzione dì ben 288,9 milioni di euro (vale a dire il 16,8 per cento che si aggiunge alla riduzione di 20,4 milioni di euro prevista dalla scorsa legge di bilancio e al decremento di 318,8 milioni di euro previsto dalla legge di bilancio 2009. L'incidenza percentuale sul totale generale del bilancio dello Stato è scesa dallo 0,28 per cento del 2008 allo 0,16 per cento di quest'anno. Non sappiamo come saranno impiegati gli 80 milioni di euro per i Beni culturali e i 7 milioni per le istituzioni culturali. Mi auguro che vengano utilizzati per ridare fiato a istituzioni prestigiose finora abbandonate a se stesse e per dare più forza alle soprintendenze mettendole nelle condizioni di continuare ad esercitare quelle funzioni di tutela previste dall'articolo 9 della nostra Costituzione e che sempre più difficilmente riescono a svolgere per la carenza di risorse umane ed economiche. Segnalo che tra le voci più penalizzate dai tagli vi è anche quella relativa alla «tutela dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria». Ne pagano le conseguenze le biblioteche nazionali di Firenze e Roma, gli archivi storici, i comitati per le celebrazioni, che sono rimasti senza risorse, gli istituti culturali inseriti nella tabella triennale della legge n. 534 del 1996, che come è noto sono in grande sofferenza, mentre altri prestigiosi enti vigilati dal MIBAC ricevono briciole o niente.

ricorrere all'aumento della benzina, proprio in questo momento di turbolenza internazionale, che ha già prodotto sensibili aumenti negli ultimi mesi. Proprio in ragione di ciò, la stessa Commissione industria invita a trovare coperture alternative a quella prevista dal Governo. Era un errore l'aumento di un euro del biglietto delle sale cinematografiche, previsto dal decreto-legge milleproroghe per rifinanziare il *tax credit* a favore del cinema e ora cancellato - ed è un errore l'incremento dell'aliquota dell'accisa su benzina e gasolio, peraltro già deciso dal direttore dell'Agenzia delle dogane.

rincaro destinato ad incidere sui prezzi, ad aumentare la pressione fiscale, a gravare sui cittadini che usano l'auto per lavoro o per necessità. Sono costi che ricadono sulle famiglie e sui consumi. evidente, poi, che entrambe le soluzioni di copertura mettono in moto un meccanismo di conflittualità con l'opinione pubblica. Danno l'idea che la cultura sia un lusso, che deve gravare direttamente sui cittadini con un di più da pagare direttamente; che essa non è affare che riguardi lo Stato. Altre soluzioni erano e sono possibili, come noi indichiamo nei nostri emendamenti, considerato che non si tratta di grandi cifre. Ci auguriamo che il Governo voglia davvero prenderle in considerazione. L'articolo 2 riguarda poi interventi di tutela dell'area archeologica di Pompei. Era ora che anche il Governo prendesse atto della necessità di interventi urgenti anziché tendere a minimizzare, come è accaduto finora con l'ex ministro Bondi. I cinque crolli che si sono succeduti in poche settimane, nei mesi di novembre e dicembre dello scorso anno, soprattutto della «*Domus* dei Gladiatori» e della «Casa del Moralista», hanno dato il segnale che si stava toccando un punto di non ritorno. Il sito di Pompei, come tutti sanno (ma è bene ricordarlo), è l'area archeologica più vasta e nota nel mondo, il secondo fra i musei italiani più visitati, con più di due milioni di visitatori l'anno: dovrebbe essere nel cuore e nella mente di chiunque governi. Così non è stato nei tre anni di questo Governo, che ha pensato bene di commissariare la soprintendenza, nominando fra l'altro non un esperto, ma un dirigente della protezione civile senza alcuna competenza in materia. Pompei ha bisogno di opere di consolidamento, di manutenzione e restauro, e non si possono certo espropriare gli archeologi della gestione di un luogo così complesso. Averlo fatto si è rivelato com'era prevedibile un errore, e lo dimostra il ricorso a mezzi impropri per un sito archeologico, come ruspe e gru, che hanno provocato, come sembra, il crollo della «*Domus* dei Casti Amanti». Le scelte da fare sono certamente impegnative: occorre dotare quel sito delle necessarie risorse umane ed economiche e di strumenti per poter garantire innanzitutto gli interventi urgenti di messa in sicurezza degli edifici più a rischio, l'immediato avvio di un adeguato piano di manutenzione ordinaria dell'intero sito ed un programma di interventi a medio e lungo termine, che rispondano alle reali esigenze di conservazione. Solo in parte però le misure previste nel provvedimento rispondono a tali esigenze; alcune di esse presentano aspetti che non ci convincono, e che vogliamo esplicitare. È noto che la soprintendenza per i beni archeologici di Napoli e Pompei gode di uno *status* speciale che le conferisce anche una speciale autonomia. Invece, già nel comma 1, a proposito della definizione di un programma straordinario e urgente di interventi, la soprintendenza viene ad avere un ruolo secondario rispetto al direttore generale per le antichità e al Ministero. Per la copertura si fa riferimento all'utilizzo anche di Fondi per le aree sottoutilizzate (FAS) destinati alla Campania, ma senza precisarne i limiti temporali, come fa osservare anche il parere della 5a Commissione. È positiva la previsione del comma 3 circa lo sblocco delle assunzioni, in deroga alla legge n. 25 del 26 febbraio 2010, attingendo a graduatorie in corso di validità sia di personale di III area che per figure dirigenziali. Personale più giovane potrà dare il suo contributo di conoscenza ed esperienza. Dal momento, tuttavia, che non è previsto un limite di validità della norma, sarebbe opportuno prevedere la possibilità di ricorrere anche a nuovi concorsi pubblici nel caso che si esaurissero le graduatorie senza che siano stati coperti tutti i ruoli consentiti dai limiti di spesa. Molto problematico per noi è, invece, il comma 4, nel quale si prevede la possibilità per la soprintendenza di avvalersi della società ALES ai fini dell'attuazione del programma di interventi di cui al comma 1. Com'è facile immaginare, il programma di interventi in questione prevede conservazione e restauro, oltre che manutenzione: funzioni che normalmente sono svolte da personale qualificato, reclutato per concorso, previa verifica delle competenze richieste. Non ci risulta che ALES s.p.a. bandisca concorsi. Di fatto, al momento manca ogni indicazione circa le forme di reclutamento del personale, dei criteri di selezione, di contrattualizzazione o del trattamento economico del suo personale facendo, temere che tale società possa essere trasformata in una vera e propria agenzia di lavoro interinale del Ministero, attraverso la quale possono essere esternalizzate anche funzioni come la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale, che costituiscono la missione stessa MIBAC. Esiste, poi, il problema relativo al rischio dell'alterazione delle regole della concorrenza, che non può considerarsi risolto dall'inciso presente nello stesso comma 4 «nel rispetto dei principi e delle disposizioni di fonte comunitaria»; tale problema è invece divenuto tanto più grave oggi, in un panorama in cui le imprese di servizi per i beni culturali stanno affrontando, anche loro, la crisi economica. Ricordo che in diverse occasioni l'Unione europea ha segnalato come l'affidamento *in house* non possa essere in nessun caso considerato come una regola, ma solo come un'eccezione, ed ha per questo richiamato l'Italia ad una maggiore moderazione nell'uso di tale modalità. Mi pare che vi siano ragioni sufficienti per proporre la soppressione di questo comma

Riteniamo che vadano esplicitate garanzie circa il fatto che tale semplificazione non incida negativamente sulla qualità degli interventi di conservazione e restauro e non rechi danno agli edifici e alle altre strutture del sito.

Anche il comma 6 presenta elementi di problematicità, quando rinvia a interventi «ricadenti all'esterno del perimetro delle aree archeologiche» che vengono dichiarati di pubblica utilità e possono essere realizzati in deroga alle previsioni di pianificazione urbanistica vigenti. Non è chiaro che cosa si debba intendere per «esterno del perimetro delle aree archeologiche», se si tratta di area demaniale oppure no. In ogni caso, sembra eccessiva una deroga tanto ampia ai normali strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale che, va ricordato, sono anche strumenti di tutela del paesaggio e delle aree urbane. Vanno introdotte anche in questo caso Non si capisce poi la logica del comma 8 che dà al Ministro il potere, in deroga alle leggi vigenti, di trasferire risorse da una soprintendenza speciale a un'altra, indipendentemente dai bisogni di ciascuna di esse e in nome di un astratto e non meglio precisato riequilibrio finanziario fra le soprintendenze speciali ed autonome. Come si vede, e concludo, l'intero articolo 2 si compone di una lunga serie di deroghe, che dimostrano la necessità di una revisione profonda dei sistemi di spesa del Ministero, dei modi di affidamento dei lavori sui beni culturali, delle attuali regole sul blocco delle assunzioni, validi per tutte le sovrintendenze, non solo per Pompei, con le adeguate garanzie di pubblicità, imparzialità, parità di trasparenza di trattamento e proporzionalità. Non sarebbe difficile se si attribuisse alla cultura un ruolo irrinunciabile, ma così finora non è stato, con questo Governo.

se, da un lato, l'esame è stato molto approfondito, con una discussione di qualità, con un confronto autentico tra la maggioranza, l'opposizione ed il Governo, dall'altro, però, l'atteggiamento del Governo e della maggioranza, orientata a rinviare all'Aula ogni decisione specifica sugli emendamenti, non ha consentito di sviluppare la discussione in termini pienamente costruttivi.

all'accoglimento di qualche nostro emendamento ci lasciano perlomeno al momento ancora del tutto insoddisfatti, sia per la vaghezza delle affermazioni, sia perché, per quanto ci è dato di capire, si riferiscono a elementi molto specifici, e forse per alcuni aspetti anche marginali. Il mio compito in questa relazione di minoranza è quello, dopo la relazione della collega Franco, di concentrarmi sugli articoli che vanno dal 3 al 7, senza però poter omettere prima una considerazione aggiuntiva sull'incremento delle accise sulla benzina e sul gasolio. Io credo che questo fatto sia particolarmente grave, perché si inscrive non solo all'interno di un più generale incremento dei prezzi dei carburanti, per ragioni di carattere internazionale - ma non è questa la sede

prezzi dei generi di prima necessità e della benzina ha, come è evidente - lo ha sottolineato anche il Governatore della Banca d'Italia - un carattere fortemente redistributivo alla rovescia, vale a dire che grava molto di più sulle fasce medie e deboli della popolazione.

uno dei nostri emendamenti che prevede che, anziché lavorare sull'incremento delle accise, si debba lavorare invece ad una riduzione, attraverso una riassegnazione e un riuso delle auto blu, delle spese che la pubblica amministrazione sostiene in questa direzione. Sarebbe un bel segnale che noi mandiamo, che manderemmo all'opinione pubblica se potessimo dire tutti insieme che l'incremento dei fondi per il FUS proviene da una ridefinizione dell'uso delle tanto bistrattate auto blu. L'articolo 3 di questo disegno di legge di conversione prevede la proroga del divieto di incroci tra settore della stampa e settore della televisione. Anziché seguire la strada più semplice e diretta di limitarsi a prorogare al 31 dicembre 2012 il termine scaduto il 31 marzo scorso, che prevede il divieto per i soggetti che esercitano un'attività televisiva in ambito nazionale attraverso più di una rete di esercitare attività di impresa editrice di giornali, si è seguita una via più tortuosa che fa sorgere il dubbio che, invece di provvedere ad una regolamentazione di carattere generale e obiettivo, si intenda - anche in questo caso - intervenire su situazioni specifiche.

In base a quali criteri oggettivi e riscontrabili si sono stabilite queste soglie? Perché non il 9 e il 41 per cento? Perché non il 7 e il 45

L'articolo 4 ridefinisce le modalità di assegnazione dello spettro radioelettrico. Vorrei brevemente analizzare il problema sotto due punti di osservazione: quello dell'emittenza locale e quello della copertura finanziaria in esito alla gara per l'assegnazione delle frequenze. La tutela del pluralismo si declina nel sistema radiotelevisivo anche riconoscendo un adeguato spazio all'emittenza locale. Per questo motivo, la legge riconosce addirittura una riserva minima delle risorse alle TV locali almeno pari Per realizzare questa serie di condizioni, le reti nazionali hanno avuto un'allocazione su gamme di frequenza più basse; le reti locali sono quasi tutte finite su frequenze che occupano i canali dal 61 al 69, che, come è noto - questo è il punto - sono tutte oggetto di riattribuzione mediante gara in favore dei servizi delle telecomunicazioni. La norma del decreto-legge introduce, quindi, una grave sperequazione in ordine al trattamento riservato alle reti locali, che sono costrette a lasciare questa porzione di spettro radio, e a quello delle reti nazionali, la cui posizione rimane inalterata. Si lede così il principio di uguaglianza e, sostanzialmente, si alterano le condizioni di pluralismo a cui pure il digitale avrebbe dovuto tendere. Il meccanismo previsto dal decreto non solo è ingiusto, ma si presenta di complicata attuazione, anche in relazione ai tempi previsti nella legge di stabilità per l'effettuazione della gara sul dividendo esterno e sulle previsioni economiche di entrata che la stessa legge ha inteso perseguire. Arriviamo così all'altro aspetto, riguardante la copertura:

Se ciò non avvenisse, scatterebbe naturalmente la clausola di salvaguardia prevista dalla legge di stabilità attualmente in vigore. Essa prevede, infatti, che nel caso in cui ciò non si realizzi - è molto probabile che ciò non si realizzerà,

dal relatore Tancredi, che abbiamo ottenuto dal Governo anche la specifica dei tagli lineari che verrebbero applicati ai Ministeri. Ciò, naturalmente, non può però esimerci dal sottolineare la gravità di un fatto di questo genere, quale verrebbe a determinarsi se ci trovassimo di fronte al fatto si non avere nel bilancio corrente la possibilità di poter confidare sulle entrate, pari a 2,4 miliardi di euro, per quanto riguarda l'assegnazione delle frequenze. In merito a tutta la vicenda relativa all'effettiva effettuazione della gara delle frequenze radioelettriche, il Governo si è mosso - a mio giudizio - in modo approssimativo e farraginoso, determinando anche delle procedure eccessivamente complesse, che daranno luogo a contestazioni di lunga e difficile gestione. prevede la sospensione per un anno della procedura di localizzazione e realizzazione nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare. pur nella sua formulazione minimalista, rappresenta, però, la pietra tombale di una politica energetica dissennata a cui si è ispirato il Governo in questi anni: tre anni persi. Né si può pensare di continuare a restare in una sorta di limbo in cui, di certo, ci sono soltanto i costi dell'energia troppo alti (in particolare per le piccole e medie imprese), la nostra dipendenza energetica dall'estero e il vero e proprio deragliamento della politica governativa in materia di promozione delle fonti rinnovabili (come testimonia il marasma, a cui stiamo assistendo, che regna nella ridefinizione degli incentivi per queste energie). Del tutto incomprensibili sono poi le ragioni per cui dalla moratoria restano escluse le procedure per l'individuazione del sito di stoccaggio delle scorie. L'articolo 6 contiene disposizioni che riguardano gli enti del Servizio sanitario nazionale della Regione Abruzzo. Mi limito a notare, perché ci saranno su questo specifico punto interventi di altri colleghi, che la norma è sostanzialmente priva di copertura finanziaria: infatti, infatti, l'ipotizzata copertura appare un'evidente forzatura, ed è per noi del tutto inaccettabile. Veniamo ora, in conclusione, all'articolo 7: un po' il cuore di questo provvedimento; sicuramente, uno dei punti che più ha scaldato il dibattito pubblico. Ci riferiamo alle discussioni aperte in ordine al tentativo di «fermare lo straniero» sulle Alpi, di impedire scalate ostili su società italiane nazionali e di porre un freno a processi di questa natura. Ora, vorrei che questa discussione venisse, per favore e per verità delle cose, riportata con i piedi per terra. Questo articolo prevede un'integrazione dell'operatività della Cassa depositi e prestiti. Su questo punto ci sono stati pareri di numerose Commissioni

«reca eccessivi e irragionevoli margini di discrezionalità nel definire i requisiti per le tipologie di società oggetto di possibili acquisizioni da parte della Cassa depositi e prestiti e ancora, a proposito della natura non regolamentare del decreto previsto dall'articolo 7: «presenta profili di criticità, in quanto esclude le normali forme di consultazione preventiva proprie degli atti di natura normativa». Avremmo potuto come opposizione fermarci qui: era più che sufficiente per dire che l'articolo, così come è scritto, è irricevibile; bastava presentare un emendamento soppressivo, e ce la saremmo cavata alla grande. Ma non ci basta questo. Il testo, dicevo, così com'è, è irricevibile, soprattutto perché mette in mano al Governo, in particolare al Ministro dell'economia, un potere del tutto discrezionale. Immaginate - e lo dico con la franchezza che contraddistingue i nostri rapporti - che cosa potrebbe succedere in Italia se davvero venisse importato il cosiddetto modello francese, vale a dire quello del Fondo strategico di investimento. qui in Aula - che il Fond Stratégique d'Investissement francese ha fatto nel 2010 interventi su 426 società. Provate a immaginare che cosa potrebbe accadere in un Paese come il nostro se, attraverso la Cassa depositi e prestiti, il Ministero dell'economia intervenisse "direttamente" (lo dico tra Altro che colbertismo, ministro Tremonti; ho detto, con un pizzico di malizia, che questo sarebbe socialismo di Stato, e forse l'articolo 41 della Costituzione, che il Ministro vuole con tanta

Credo però che l'opposizione non possa limitarsi ad una semplice e generica polemica. Uno strumento di politica industriale (questo è quello che si propone con l'articolo 7) senza una politica industriale. allora sarebbe stato meglio ragionare prima sui punti qualificanti di una politica industriale e poi prevedere gli strumenti per applicarla. Vorrei specificare che noi non siamo pregiudizialmente contrari a dotarci di uno strumento per la politica industriale. Con altrettanta chiarezza però voglio dire che pregiudizialmente contrari non lo siamo a determinate e molto chiare condizioni: a determinate e molto chiare condizioni: in primo luogo, in un quadro, in un contesto, anche culturale, oltre che economico, di piena internazionalizzazione della nostra economia. abbiamo voluto dimostrare questo nostro orientamento esprimendolo con nostri specifici emendamenti. Ne richiamo qui soltanto alcuni.

che va incontro ad una necessità molto diffusa nell'apparato produttivo italiano, e cioè la necessità di sostenere il sistema delle piccole e medie imprese a fronte dei ritardati pagamenti della pubblica amministrazione. Per evitare il rischio, segnalato in modo puntuale dalla Ragioneria generale dello Stato, di riclassificazione del debito della Cassa depositi e prestiti come debito pubblico, nel caso in cui essa agisse per conto dello Stato nell'operazione di anticipazione dei crediti della pubblica amministrazione, noi abbiamo presentato un emendamento un po' più raffinato che prevede la costituzione di un veicolo societario specifico che va sul mercato e che può essere partecipato anche da investitori privati: un veicolo nella forma della società per azioni, che risponderebbe, come nel caso di prese di partecipazione della Cassa depositi e prestiti, solo con il proprio patrimonio e non rideterminerebbe mai, quindi, un problema di riclassificazione della Cassa depositi e prestiti all'interno del debito dello Stato. Il Governo si era «riservato», come si usa dire. Speriamo che questi giorni abbiano portato al Governo un elemento di rasserenamento su tale punto e che possa essere accolto questo che è un emendamento importante, non per l'opposizione ma per il sistema delle piccole e medie imprese.

possa assumere partecipazioni, in questo caso anche di controllo - sottolineo questo passaggio per quanto dirò successivamente - in società proprietarie di infrastrutture energetiche nazionali e sovranazionali. Il riferimento esplicito è alla separazione proprietaria di SNAM Rete Gas da ENI anche al fine della costruzione di un mercato interno realmente concorrenziale. Il secondo filone d'intervento emendativo che caratterizza i nostri emendamenti riguarda la società chiamata ad acquisire partecipazioni. Questa società, che sulla base di quanto è stato proposto nella modifica dello Statuto della Cassa depositi e prestiti dieci giorni fa dovrebbe essere un veicolo nuovo che acquisisce partecipazioni, si troverebbe ad agire su un territorio delicatissimo che è quello di confine tra pubblico e privato. Allora, è bene che in quel territorio di confine si agisca con requisiti molto chiari. luogo, requisiti di trasparenza, di grande professionalità, con partecipazioni che siano sempre di minoranza, con certezza dei tempi di dismissione, con rendicontazione al Parlamento e all'opinione pubblica di quello che si fa. La Cassa depositi e prestiti, a nostro giudizio e attraverso i nostri emendamenti, opera dunque solo attraverso quel veicolo nella presa di partecipazione, e noi auspichiamo che quel veicolo, per ragioni di trasparenza, sia appunto un veicolo quotato. Proviamo a immaginare l'ipotesi di un intervento nelle banche, che è stato escluso ‑ ne prendiamo atto ‑ ai margini dell'assemblea per la modifica dello Statuto della Cassa depositi e prestiti, ma che è ancora presente nel dibattito.

decidesse di intervenire nell'aumento di capitale di una banca nella quale le stesse fondazioni che partecipano alla Cassa depositi e prestiti sono azioniste di controllo effettivo. Saremmo davvero

sottolineando che i requisiti di comprovata professionalità e di elevata qualificazione e competenza, di indiscussa moralità e di indipendenza devono contraddistinguere i componenti del *board* e l'amministratore delegato di questa società che acquisirà le partecipazioni,

Tutto, infine, deve essere portato all'attenzione del Parlamento, anche alla luce di quanto positivamente è stato deciso ‑ voglio sottolinearlo ‑ in sede di riforma dello Statuto della Cassa depositi e prestiti, dove si prevede che la Cassa possa intervenire solo in società che siano in sostanziale equilibrio economico.

ha un drammatico bisogno di una politica capace, nell'ordine, di raggiungere questi tre obiettivi: assumere un orizzonte di medio-lungo periodo per l'adozione di scelte di finanza pubblica, sia dal lato delle uscite sia dal lato delle entrate;

senza i quali la produttività del lavoro e quella totale dei fattori continueranno a declinare, costringendoci a quella crescita incerta e stentata che dura da 15 anni e che si è interrotta nel corso del 2008 e del 2009 solo per dare luogo alla più pesante caduta del prodotto che la grande recessione abbia provocato nei maggiori Paesi europei; nei maggiori Paesi europei; realizzare o, meglio, favorire con l'attività regolatoria la realizzazione di infrastrutture materiali e immateriali, che reclamano investimenti a redditività molto differita nel tempo. Le grandi reti di telecomunicazioni e dell'energia sono in questo contesto l'esempio più immediato, poiché sono la sede, per parafrasare il vecchio Carlo Marx, dell'accumulazione nell'epoca del capitalismo postfordista. dunque programmazione di medio periodo, più investimenti diretti esteri, regole certe per le infrastrutture delle grandi reti. grandi reti. Colleghi della maggioranza e del Governo, se vogliamo una rappresentazione quasi fisica del drammatico *deficit* di efficacia della politica italiana in generale (vi comprendo l'opposizione), e del Governo in particolare, dobbiamo leggere in sequenza i pochi articoli di questo decreto. (si badi, non la rimodulazione, l'aumento o la diminuzione: l'abrogazione) del prelievo di un euro stabilito dalla legge n. 10 del - attenzione alla data - 26 febbraio 2011 su ogni biglietto del cinema, sostituendone integralmente il gettito con un aumento dell'accisa sulla benzina e sul gasolio da autotrazione. Dunque, il 26 febbraio di quest'anno si compie una scelta, bella o brutta che sia, a forte impatto su un settore rilevante della nostra industria culturale, come è l'attività cinematografica. Dopo 33 giorni la si toglie di mezzo e si dispone un aumento di quella che è l'odierna versione della tassa sul macinato di un tempo, cioè l'accisa sulla benzina. Cosa è accaduto, colleghi della maggioranza, colleghi del Governo, in questi 33 giorni a motivare una scelta tanto contraddittoria? Nel settore del cinema una cosa è accaduta: se ne è andato il ministro Bondi; nel settore dell'energia si è accentuata la corsa all'aumento del prezzo del petrolio; nell'economia, di conseguenza, si sono riaccesi preoccupanti fuochi di inflazione, tanto da indurre la BCE ad alzare il tasso di riferimento proprio la settimana scorsa. Lasciamo stare - per bontà d'animo non si infierisce - il trattamento così riservato dalla maggioranza e dal Governo al ministro Bondi, e occupiamoci del resto. Disponendo l'aumento dell'accisa sulla benzina per coprire una nuova spesa, il Governo e la maggioranza compiono due scelte gravissime: contravvengono in modo clamoroso, patente, esplicito, senza nemmeno cercare di nascondere la sostanza, ad una regola ormai implicita ma fondamentale della legge di contabilità, che vieta in corso d'anno di coprire nuova spesa con l'aumento della pressione fiscale; in secondo luogo, gettano benzina - in senso proprio, in questo caso - sul fuoco dell'inflazione, che infatti sta robustamente rinvigorendosi, crescendo in Italia, il Paese in cui la ripresa è più debole, per cui dovremmo attenderci,

Altro che programmazione di medio-lungo periodo, dunque; il Governo vive e decide giorno per giorno, ora prende, ora toglie, senza alcuna strategia, senza alcuna razionale motivazione. Va avanti, come dicono Berlusconi e Bossi: sì, va avanti, ma non sa verso dove. sa verso dove. Siccome non vogliamo mai fare solo una valutazione critica, su questo primo punto, e limitatamente a questo decreto, si può porre rimedio? Certamente sì, e lo abbiamo inutilmente proposto: via l'aumento dell'accisa, rimangiatevelo, perché è una scelta irresponsabile; finanziamo il FUS con una drastica riduzione della spesa oppure - e per noi è una subordinata, lo sottolineo - istituite, se proprio volete coprire con un aumento

le cose - se possibile - vanno ancora peggio, anche se peggio di così è difficile. In un Paese nel quale la quota di aziende situate sul territorio nazionale e controllate da capitali esteri è la più bassa d'Europa tra i grandi Paesi (il 4,1 per cento in Italia contro la la Francia statalista che ha il 10,3 per cento di aziende situate in Francia che sono di capitale estero, più del doppio dell'Italia, e il 12,2 per cento nel Regno Unito, ma quello è il capitalismo anglosassone, tanto odiato: non parliamone nemmeno, ci mancherebbe), ci mancherebbe), in un Paese così, dove non ci sono investimenti esteri, dove non siamo capaci di attrarre investimenti, adottiamo per decreto una norma che autorizza (leggete quella dell'articolo 7, perché la gente non ci crede; quando dico che c'è un decreto, una legge dello Stato, una norma che dice questo, non ci crede nessuno: bisogna che vada in giro con l'articolo, altrimenti non ci credono) credono) lo Stato italiano, tramite la controllata Cassa depositi e prestiti, a comprarsi le società che crede o, meglio, le società che il Ministro dell'economia, a suo totale arbitrio e senza nemmeno far passare il decreto nel Consiglio dei ministri o in Parlamento, crede di voler acquistare.

dell'intervento su operazioni davvero strategiche, come ad esempio una grande società unitaria delle reti energetiche gas ed elettricità, per realizzare un grande *player* di un mercato dell'energia europeo da unificare costruendo le infrastrutture di interconnessione. Avete detto no a tutto, signor Sottosegretario, per difendere l'italianità delle imprese. Non prendiamoci in giro: l'unica cosa che viene difesa con operazioni di questo tipo - come è dimostrato da tutti i precedenti - è l'attuale assetto del capitalismo italiano, blindato dentro patti di sindacato tanto impenetrabili quanto asfittici. Per questo motivo, i capitalisti che stanno dentro il patto di sindacato e vogliono difendere le loro posizioni sono ben disposti ad accettare

riguarda le grandi infrastrutture, vengono al pettine i nodi della gestione delle frequenze liberate dal passaggio al digitale terrestre; di nuovo, siamo alla prova provata della totale mancanza di visione del Governo.

cioè un insieme di frequenze, a RAI e Mediaset, quando avrebbe potuto assegnarne loro almeno un terzo di meno senza alcun danno per i nostri beneamati, rispettivamente, duopolisti.

megahertz; qualche giorno dopo avere compiuto questa brillante scelta, quasi inconsapevole di sé, con la legge di stabilità ha disposto che quelle stesse frequenze, che aveva appena finito di regalare, siano oggetto di una gara con l'obiettivo di far entrare nel bilancio dello Stato entro e non oltre il 30 settembre di quest'anno almeno 2,4 miliardi di euro.

con il rischio serissimo che la gara non possa espletarsi nei tempi previsti. Ciò ha due conseguenze gravissime. La prima è che gli investimenti delle TelCo, delle grandi compagnie di telecomunicazioni, per l'utilizzazione delle nuove frequenze non si realizzino nei tempi previsti, ed il Paese quindi resti privo di una infrastruttura essenziale per la sua modernizzazione e la sua capacità competitiva; continuiamo a blaterare di banda larga,

è che scatti la clausola di salvaguardia prevista dalla vigente legge di stabilità e gli accantonamenti diventino tagli a tutti i Ministeri, per una somma pari a 2,4 miliardi di euro.

ma in questa sede ogni volta assistiamo a delle sceneggiate che considero invereconde sulla storia della benzina delle auto dei carabinieri e della polizia. Vi informo

Tutto ciò senza alcun criterio, perché se si fanno tagli in quel modo, non c'è criterio che non sia quello di fare in modo che il totale dia 2,4 miliardi. L'unico criterio è questo: tutti gli altri sono banditi, non si possono nemmeno considerare. si possono nemmeno considerare. Si può ancora evitare questa catastrofe? Forse sì, anche se è più difficile che nel caso precedente: bisogna creare le condizioni perché la gara si possa svolgere nei tempi fissati dalla legge di stabilità. C'è un solo modo per farlo: meno frequenze alla RAI e Mediaset (almeno un terzo bisogna togliergliele) e un po' di soldi in più di quelli previsti alle se, questi ultimi soldi, diciamo la verità, bisognerebbe farli pagare personalmente, come risarcimento per danno erariale, a chi quelle frequenze le ha concesse gratuitamente o quasi alle ancora nel settembre scorso e ora vorrebbe riacquistarle con i soldi dei contribuenti. Signor Presidente, onorevoli rappresentanti del Governo, colleghi, le misure contenute nel provvedimento in esame sono senz'altro di grande rilievo, soprattutto per quanto concerne i settori di competenza della 7a Commissione. Va dato atto al Governo di aver corrisposto finalmente alle grandi attese del mondo della cultura, che a più riprese, anche con manifestazioni di protesta, aveva sollecitato un reintegro di fondi. L'Esecutivo ha dunque agito al massimo delle possibilità nel momento in cui le risorse si sono rese disponibili. Certo, è innegabile che, rispetto ai *desiderata* degli operatori del settore, si renderanno necessarie ulteriori misure di sostegno; questo spiega del resto le proposte emendative presentate, alcune anche a mia firma, che tentano di ovviare ad altre problematiche irrisolte, soprattutto in termini finanziari. Cito, ad esempio, la possibilità di rimpinguare gli stanziamenti di altri enti, anch'essi di primaria importanza, come il Museo della scienza e della tecnica di Milano, per il quale ho previsto, insieme al senatore Giancarlo Serafini, la destinazione di due milioni di euro nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 1. L'orientamento prevalente nella sede di merito è stato tuttavia quello di attenersi all'oggetto specifico del decreto: dunque non è stato possibile introdurre altre forme di intervento per i beni culturali, che alleggerissero per gli stessi il peso della manovra estiva dello scorso luglio. Mi riferisco in particolare alla possibilità di escludere gli enti culturali dal taglio delle spese per convegni e mostre, per sponsorizzazioni,

i contenuti di un disegno di legge presentato in Senato a prima firma del senatore Cursi in materia di piccole e medie imprese di spettacolo, che avrebbe consentito l'estensione a queste ultime delle agevolazioni nazionali e comunitarie previste dalla normativa vigente per le piccole e medie imprese. Ciò avrebbe senz'altro facilitato l'azione di tutti quei soggetti che a vario titolo operano nel comparto, cui va senz'altro riconosciuta la forma giuridica di impresa dato il ritorno economico che la loro attività determina sul mercato; non volerlo recepirelo considero un errore non di poco conto. Riconosco tuttavia che misure siffatte richiederebbero forse un provvedimento diverso e dunque, in tale logica, non è possibile allo stato un loro inserimento nel decreto, di fatto assai limitato nel contenuto. Ritengo comunque opportuno riportare l'attenzione dell'Aula sull'importanza di intervenire in ambiti che sembrano avere a prima vista un minor impatto sull'economia del Paese, ma che invece ne connotano tanto il sostrato culturale quanto proprio il tessuto economico. Alla cultura infatti non può non riconoscersi anche l'importante ruolo di rappresentare il Paese all'estero, e soprattutto essa può costituire una grande risorsa per rilanciare l'economia. La scelta qualificante di questo Governo è però quella di favorire interventi che puntino all'efficienza e che dunque presuppongano preventive riorganizzazioni, nell'ottica di allocare la spesa in maniera razionale. La natura economica del provvedimento è basata su questo presupposto, e dunque in un quadro siffatto si inseriscono pienamente gli articoli 1 e 2. Mi auguro soltanto che si possa trovare presto nuovo spazio anche per norme non esclusivamente di natura finanziaria. La discussione nelle Commissioni riunite ha del resto dimostrato la piena capacità del Parlamento di confrontarsi in maniera approfondita sui grandi temi strategici del Paese, superando posizioni preconcette, alla ricerca di soluzioni concrete. Credo che il numero relativamente basso di emendamenti presentati e la serenità del dibattito fino ad ora svolto siano una prova tangibile di ciò, cui però deve corrispondere un orientamento preciso dell'Esecutivo, soprattutto in risposta ai quesiti e alle alternative che sono emerse dall'attività emendativa circa i diversi contenuti del decreto. In questo si sostanzia, di fatto, il rapporto tra il testo presentato dal Governo e le proposte di iniziativa parlamentare, dal quale potrà emergere l'apertura necessaria per eventuali riformulazioni, rispetto alle quali, peraltro, nelle Commissioni riunite è emersa una certa disponibilità da parte dei relatori e del Governo. Sono certo che il testo che sarà licenziato dall'Aula terrà conto del contributo di tutti. *(Applausi dal Signor Presidente, ringrazio i relatori di maggioranza e di opposizione. Oggi siamo chiamati a discutere e ad approvare questo decreto *omnibus*. Si tratta di un maxicontenitore di tante disposizioni - come hanno ricordato i colleghi - frutto di una tecnica legislativa

È vero che le emergenze vanno affrontate, ma se ci fosse una programmazione più razionale e più ponderata, sicuramente non ci troveremmo oggi a dover affrontare la Così siamo chiamati ad approvare 7 diversi articoli, che spaziano - lasciatemi usare questa espressione - con incredibile naturalezza dal reintegro del Fondo unico per lo spettacolo alla moratoria sul nucleare (cito solo questi, in quanto i miei colleghi li hanno analizzati e sviluppati nella loro interezza: tante disposizioni che producono in maniera esponenziale altrettanto perplessità). Per esigenze di tempo, mi soffermerò solo su alcune norme. Parto dall'articolo 1 di questo decreto, che prevede un finanziamento

di 50 milioni di euro per ciascun anno, dal 2011 al 2013, il capitolo di bilancio relativo alla tutela e valorizzazione dei beni culturali. Ricordo che Federculture, all'indomani della manovra estiva, aveva lanciato l'allarme sul rischio paralisi del settore, denunciando che i tagli inferti finivano con il compromettere la nostra cultura, le nostre città d'arte, i nostri musei, la musica, il cinema e tutto ciò che l'Italia oggi fortunatamente detiene. Quindi, il Governo fa un dietrofront coglie l'occasione per cancellare dal mondo giuridico quella infelice disposizione del milleproroghe che aumentava di un euro il costo del biglietto del cinema; un aumento che rischiava di

Come sappiamo, però, tutto ha un prezzo e il costo di questo ravvedimento operoso si realizza con l'aumento delle accise sulla benzina. A pagarne le conseguenze saranno tutti i cittadini e - secondo stime accreditate - quest'anno un pieno di benzina costerà dai 36 ai 44

Ricordo a tutti che proprio in quest'Aula, mercoledì scorso, il ministro per i beni e le attività culturali Galan, da poco nominato, usando una espressione in verità poco felice e poco adatta al mondo culturale, ha affermato che la cultura è la benzina del Paese. A questo punto abbasso il tono di voce perché mi vergogno a dover dire che è chiaro per quale motivo il Governo in questo decreto inserisce proprio una tassa sulla benzina: sembra che ci sia una schizofrenia governativa e non una programmazione governativa. Non illudiamoci, però, che questo provvedimento possa segnare un effettivo rilancio del comparto cultura. Infatti, il Governo non ha speso una parola su come mettere in campo ‑ per esempio ‑ grandi figure professionali e manageriali in grado di far crescere il nostro panorama culturale, per renderlo realmente un motore importante della nostra economia. L'Italia possiede le stesse ricchezze culturali degli altri Paesi, anzi ne possiede anche di più in termini qualitativi e quantitativi. Per esempio, andare agli Uffizi di Firenze e vedere «La Primavera» di Botticelli, oppure innamorarsi del sorriso della Gioconda al Louvre di Parigi, o ancora, ammirare la Stele di Rosetta al British Museum di Londra ci danno la misura di quanto il nostro Paese sia culturalmente alla pari, per non dire superiore. Peccato che, mentre il Louvre ha una buona gestione finanziaria, quella dei nostri musei lascia purtroppo a desiderare, perché mancano e vengono continuamente decurtati i fondi pubblici. pubblici. Da un Presidente imprenditore ci saremmo aspettati una gestione manageriale dei nostri giacimenti culturali, che lui potrebbe definire - se il ministro Galan li ha definiti la benzina del Paese - il petrolio del nostro Paese, un patrimonio quindi che dovrebbe essere raffinato e reso produttivo, ma di fatto non si fa nulla non si fa nulla di questo. Infatti, ad oggi, se si assumesse il RAC, che è un indicatore economico sintetico, per esprimere la valorizzazione dei musei, dando all'Italia un valore pari a 100, quello della Francia sarebbe pari a 400 e quello del Regno Unito raggiungerebbe i 600. i 600. Secondo ricerche dello stesso Ministero per i beni e le attività culturali, solo un centinaio dei nostri musei è dotato di un servizio di *merchandising* ben organizzato, senza considerare che i fondi per la cultura che l'Europa attualmente eroga restano non investiti proprio a causa dell'assenza di figure specifiche che facciano da mediatori tra i nostri enti locali e l'Europa. Con un intervento serio, mutuando l'esperienza consolidata degli altri Paesi, gli Uffizi non raccoglierebbero più solo 1,6 milioni di visitatori l'anno, ma potrebbero arrivare agli 8,5 milioni del Louvre, o forse È dunque sotto gli occhi di tutto il collasso del comparto cultura, un settore strategico per l'intera economia del Paese, che non viene adeguatamente valorizzato e finanziato.

apposito emendamento, che si spera possa essere approvato. Inoltre, sarebbe stato certamente risolutivo riconoscere ai lavoratori del settore le provvidenze legislative in materia di ammortizzatori sociali e gli strumenti per il sostegno del reddito. Prima la collega Franco Vittoria ha ben sviscerato

Proprio il ministro Galan, il 13 aprile scorso, ha sottolineato che «investire nel settore della cultura non è indispensabile ma fondamentale» ed ha invitato tutti, a prescindere dalle appartenenze politiche, a cooperare in iniziative volte alla promozione del comparto.

questa sede quanto è stato finora fatto, senza considerare che l'appello del Ministro al coinvolgimento degli enti locali nel rilancio della cultura rischia di rimanere lettera morta dato il divieto, oggi operante per le pubblica amministrazioni, di effettuare spese per mostre e pubblicità.

il Governo, perde una buona occasione per segnare un effettivo cambio di rotta nella gestione della politica economica e culturale del Paese, lanciando peraltro all'opinione pubblica il messaggio per cui la cultura

vorrei citare un passo tratto dal «*De re publica*» di Cicerone, secondo cui in politica «Un solo proposito tutti devono nutrire, che il vantaggio del singolo si identifichi con quello comune, poiché se uno lo assume egoisticamente per sé ogni umano consorzio ritiene dissolto». Credo che oggi ci sia davvero bisogno di ricordare questo insegnamento di Cicerone e far sì che la politica

questo decreto-legge provvede a incrementare, a decorrere dall'anno 2011, la dotazione del Fondo unico per lo spettacolo (FUS), a sostenere spese per la manutenzione e conservazione dei beni culturali e per interventi a favore di enti ed istituzioni culturali; prevede una serie di iniziative a favore della Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e Pompei; proroga al 2012 il divieto di incroci tra giornali e TV; stabilisce il calendario definitivo per la transizione alla alla trasmissione televisiva digitale terrestre; stabilisce infine alcune disposizioni speciali per la Regione Abruzzo. Desidero soffermarmi solo su alcuni aspetti. Il programma Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo con uno stanziamento in conto competenza pari a 298,6 milioni di euro per il 2011, ha subito una riduzione di circa 153,3 milioni di euro rispetto al dato assestato del 2010,

potrebbe determinare di fatto la chiusura di interi settori di attività che, al contrario, sono da considerare strategici per il Paese e necessitano di progettualità, sia in termini di finanziamento che di programmazione e di politica di interventi. Nel programma rientrano, in particolare, gli stanziamenti per il Fondo unico per lo spettacolo, con 258,6 milioni di euro (meno 36 per cento rispetto al dato assestato 2010, pari a 414,6 milioni di euro). Esprimo soddisfazione per il sostegno che il Governo intende dare alle fondazioni lirico sinfoniche, che la riduzione degli stanziamenti destinati alla cultura aveva messo in grave sofferenza. Il Governo ha previsto nel decreto‑legge cosiddetto milleproroghe norme di rifinanziamento per il 2011 di tali fondazioni, per un importo pari a 15 milioni di euro quale apposita integrazione del FUS, con l'esclusione di alcune specifiche fondazioni cui è destinato un importo di tre milioni di euro ciascuna (Arena di Verona, Teatro La Scala di Milano). La normativa previgente in materia ha evidenziato alcuni elementi di criticità, che non hanno permesso di raggiungere gli obiettivi prefissati dal legislatore. È infatti venuto meno il presupposto base del decreto legislativo n. 367 del 1996, la centralità del finanziamento pubblico, che ha seguito l'andamento decrescente del Fondo unico per lo spettacolo, senza che a ciò corrispondesse un'adeguata incentivazione della partecipazione dei privati attraverso la defiscalizzazione del loro contributo. A ciò va aggiunto che la normativa successiva al citato decreto ha fatto cadere alcuni requisiti imprescindibili nella trasformazione degli enti in fondazioni, quali l'apporto dei privati e l'equilibrio economico finanziario tra pubblico e privato, provocando forzate trasformazioni. La razionalizzazione dell'intervento pubblico e l'incentivazione del finanziamento privato in campo culturale restano quindi ancora al centro di ogni processo riformatore nell'ambito della cultura e dello spettacolo. razionalizzazione, nel prossimo futuro, dovrà prevedere una serie di azioni quali, innanzitutto, interventi sulla *governance* delle fondazioni lirico-sinfoniche, attraverso la rivalutazione dei legami con il territorio. La riforma attuata non ha, a mio avviso, inquadrato correttamente il ruolo dei Comuni: sarebbe stato più opportuno collocare la riforma approvata nella visione federalista, in modo da assicurare un bilanciamento tra intervento centrale e autonomie. la revisione dei criteri di finanziamento, valorizzando la progettualità e l'identità delle singole istituzioni. Il contributo dello Stato è insostituibile, purché si raggiunga un equilibrio tra i finanziamenti statali, degli enti locali e dei privati da un lato e i ricavi ottenuti dalla vendita dei biglietti dall'altro. Attualmente, a fronte di un'assenza quasi totale di *sponsor* privati e di entrate irrisorie, la maggior parte delle risorse è di fonte statale, a dispetto della natura giuridica delle fondazioni. Anche per quanto riguarda il cinema, il contributo statale non può più seguire i percorsi automatici, ma deve essere mirato a sostenere i giovani, la sperimentazione e l'innovazione. La disciplina vigente, frutto della riforma del ministro Urbani di sei anni fa, ha avuto il merito di dettare regole di trasparenza e di efficienza, eliminando aree di eccessiva discrezionalità, ridisegnando i meccanismi di riconoscimento dei benefici, ponendo termine a decennali sprechi di risorse e dando luogo ad una prima fase di risanamento, coincisa non a caso con il quadriennio di rinascita, di affermazione, nel Paese e all'estero, del cinema italiano di qualità. Il contesto attuale, caratterizzato dalle ricadute negative di una crisi economica generale che ha imposto tagli dolorosi ma inevitabili, non appare essere tra i più favorevoli all'introduzione di una nuova riforma di sistema del sostegno pubblico all'attività cinematografica. La risposta risiede ancora una volta nella defiscalizzazione e nel federalismo economico; quindi la gestione dei fondi dovrebbe essere delegata alle Regioni, e ciò per un principio di sussidiarietà e di eterogeneità delle diverse realtà. *(Applausi

di un Governo privo di bussola, che sforna decreti estemporanei, misure tampone in assenza di una strategia di lungo periodo per far uscire il Paese dalla crisi sistemica ed agganciare la crescita economica che non c'è. Ho già avuto modo di esprimere in Commissione le criticità sulla finta moratoria in merito all'opzione sul nucleare, che dopo l'incidente di Fukushima, peggio del disastro di Chernobyl, bisognerebbe abbandonare definitivamente. Egualmente abbiamo criticato i rapporti incestuosi tra settori della stampa e della televisione, assieme alla mancata razionalizzazione dello spettro radioelettrico. che voglio sviluppare riguarda due temi cari ai consumatori ed ai risparmiatori, soprattutto oggi che il tribunale di Milano ha assolto le banche sul *crack* Parmalat, quasi che i risparmiatori se la fossero andata a cercare. Le questioni che ci interessano riguardano la gestione della Cassa depositi e prestiti, destinata a sostituire il "lattaio di Collecchio" con criteri così oscuri e discrezionali da aver suscitato anche i distinguo della Commissione affari costituzionali; la guerra tra i poveri, che questo Governo è aduso ad alimentare, con la tassa sul cinema che sarà pagata dai consumatori due volte, sia con l'incremento delle accise sulla benzine, che con il conseguente aumento dell'inflazione.

Voglio anche ricordare che proprio in questi giorni la Banca centrale europea ha eseguito la prima manovra, delle tre previste, di incremento del costo del denaro, dovrebbe portare il tasso di riferimento dall'1 all'1,75, e addirittura al 2 per cento nel 2011, con ricadute da 140 fino a 200 euro per 3,2 milioni di mutuatari indebitati a tasso variabile, che hanno seguito i cattivi consigli delle banche.

soia ed altre *commodities*), omettendo di fare i nomi degli speculatori, che sono i suoi amici banchieri della Goldman Sachs e di altre banche di affari, che hanno scatenato la rivolta del pane in Nord Africa. E, di fronte a questo, il Governo non trova di meglio che far gravare sui consumatori il finanziamento della cultura, in una partita di giro, che il ministro Tremonti in passato avrebbe definito di raggiro. Ci saranno gravi conseguenze per le tasche dei cittadini che, oltre ai profitti della filiera petrolifera, alimenteranno anche le casse dello Stato. Voglio ricordare che, rispetto allo scorso marzo, l'IVA - tassa mobile al 20 la benzina di 4 centesimi al litro, e di altrettanto per il gasolio. Voglio ricordare che l'erogazione dei carburanti è stimata in miliardi di litri, e su questi si applicano gli aumenti di IVA:

che finanzia la cultura! Se a ciò poi aggiungiamo gli ulteriori aumenti decisi sull'accisa della benzina di 2 centesimi al litro, il ricavo complessivo raggiungerà la cifra di 2.124 milioni di euro. Tali aumenti dei carburanti incidono sulle famiglie italiane per costi diretti di 240 euro in più all'anno, a cui si aggiungono ricadute di 170 euro per i costi indiretti, dovute al fatto che buona parte dei beni è trasportata su gomma, per un totale di 410 euro. E questo sarebbe un Governo che non mette le mani nelle tasche degli italiani! Invece di verificare la doppia velocità dei prezzi dei carburanti, l'apertura della vendita attraverso la grande distribuzione, un blocco settimanale degli aumenti, un acquirente unico che potrebbe calmierare i prezzi, la liberalizzazione (dato che le cosiddette pompe bianche, non obbligate ad acquistare dalle «sette sorelle», riescono a praticare prezzi con sconti anche di 10 centesimi al litro), il Governo mette le mani nelle tasche degli italiani.

Su queste accise viene applicata anche l'IVA, una tassa sulla tassa. Il Governo non interviene per far abbassare i prezzi dei carburanti, perché più essi sono elevati più lo Stato, che diventa l'«ottava sorella», ci guadagna, quanto la tassazione non comprende solo l'accisa ma anche l'IVA. Il decreto che consente alla Cassa depositi e prestiti di poter utilizzare risorse provenienti dalla raccolta postale per interventi a difesa dell'italianità - abbiamo visto Lactalis e altro ancora - riguarda anche Bondi. Mi riferisco al commissario strapagato di Parmalat, che, invece di utilizzare 1,5 miliardi di euro di risorse finanziarie accumulate per rafforzare la posizione di mercato e la capacità di resistere ai tentativi di scalata, ha accumulato un tesoretto che fa gola agli scalatori. Voglio augurarmi che la difesa dell'italianità di Parmalat non possa replicare quanto accaduto con Alitalia, data l'identità dei protagonisti capeggiati da Banca Intesa, che hanno addossato alla fiscalità generale oneri per 3 miliardi di euro, a favore dei soliti «capitani coraggiosi»: Passera, Sabelli e Colaninno. e Colaninno. In merito all'individuazione dei requisiti, anche quantitativi, delle società che potranno essere acquistate da Cassa depositi e prestiti, demandata a un successivo regolamento del Ministro dell'economia, mi limito a ribadire che, come nel caso della Protezione civile gestita da Bertolaso, discrezionalità e opacità sono nemiche della trasparenza necessaria al buon andamento delle pubbliche amministrazioni per prevenire i diffusi fenomeni fraudolenti.

nel definire i requisiti per le tipologie di società oggetto di possibili acquisizioni da parte della Cassa depositi e prestiti S.p.A.». Altro che colbertismo, signor Presidente: ci avviciniamo al socialismo irreale! *(Applausi

Ho sentito dire che i crolli nel sito archeologico sono da ascrivere all'impreparazione del commissario e, implicitamente, all'*ex* ministro Bondi, che lo ha nominato. Vorrei sottolineare che in Campania questo è stato l'anno più piovoso degli ultimi 100 e che a Pompei vi sono ben 90 chilometri di muretti a secco, perché la malta di 2.000 anni fa non c'è più. Inoltre, i crolli si sono registrati tutti a ridosso del terrapieno che delimita Via dell'Abbondanza, che non è scavato pieno di terra e lapilli si gonfia con l'acqua come una spugna e preme sui vecchi muri, facendoli crollare. È il caso della «*Domus* dei Gladiatori», che oltretutto aveva un lastrico pesantissimo in cemento armato (il restauro è degli anni '50); una mostruosità archeologica, pericolosa - soprattutto il lastrico - per la stabilità della costruzione antica. Lo stesso dicasi per la «Casa del Moralista», che si trova a ridosso del terrapieno non scavato e gonfio d'acqua.

puntualizzare solo questi due aspetti. Vorrei anche aggiungere che il nuovo ministro Galan, parlando a Pompei la settimana scorsa, ha sottolineato che, date le condizioni

con questo intervento intendo rivolgermi espressamente alla Presidenza, e in particolare al Presidente del Senato. Questa legislatura non si è certo distinta per il rispetto delle procedure ordinarie di formazione delle leggi. Frequenti sono state infatti, come ben sappiamo, le deroghe sotto forma di decretazione di urgenza e, in esse, la pratica dei decreti *omnibus* o il ricorso sistematico alla fiducia. Abbiamo assistito insomma, e purtroppo la sensazione è che assisteremo ancora, ad una ricorrente pratica di delegittimazione della essenziale prerogativa parlamentare. Molteplici sono stati in questi anni e in misura crescente i richiami che il Presidente della Repubblica ha eccepito sulla decretazione con riguardo alla costituzionale: alcuni accettati dal Governo (è sembrato a malincuore), altri lasciati cadere. Nessuna illusione pertanto mi faccio sulla reale possibilità che questo mio appello alla sensibilità della Presidenza del Senato possa avere successo di ascolto e di conseguenze. nonostante, ritengo ugualmente doveroso formulare alcuni rilievi, apparentemente irrilevanti, ma a mio avviso anche essi sintomo di un evidente clima di generale diffusa disattenzione al rispetto sostanziale delle procedure. Mi riferisco, nell'ambito delle procedure interne alla nostra Camera, a quelle di assegnazione dei provvedimenti alle Commissioni indicate come referenti per l'Aula. Abbiamo assistito come membri dell'8a Commissione, nel corso di questa legislatura, ad una reiterata esclusione della Commissione dai provvedimenti che più da vicino riguardavano le nostre competenze. Ciò è avvenuto quando, in particolar modo, la decretazione *omnibus* del Governo ha costretto la Presidenza delle due Camere a scegliere secondo il criterio di competenza prevalente l'attribuzione del provvedimento alle Commissioni referenti per l'Aula, cosa avvenuta in termini inevitabilmente discrezionali. Ad aggravare la sensazione di frustrazione, si è poi talvolta aggiunto il fatto che l'argomento del provvedimento in questione era stato precedentemente oggetto da parte della 8a Commissione di indagini conoscitive o di specifici lavori di approfondimento o, ancora, di elaborazione di pareri su decreti legislativi del Governo. Ricordo che è stato così per il trasporto universale ferroviario, in occasione dell'esame del decreto in materia di interventi urgenti di revisione dei prezzi, o per le norme sull'autotrasporto, in occasione dell'esame del milleproroghe, o ancora, come nel caso in questione, per le rilevanti norme di modifica al codice degli appalti (commi 5 e 7 dell'articolo 2), piuttosto che per l'assegnazione delle frequenze radioelettriche (articolo 4).

Anche oggi è questa l'anomalia che registriamo, che sarà peraltro reiterata anche su un analogo provvedimento riguardante lo statuto delle imprese, attualmente all'esame della Commissione industria. Sarebbe stato utile per l'Aula giovarsi delle competenze dell'8a Commissione nell'esame dei provvedimenti che ineriscono materie di specifica competenza. Pertanto, in queste ricorrenti circostanze la Presidenza potrebbe avanzare un autorevole richiamo al Governo affinché si attenga ad una decretazione più omogenea prevedendo, come per l'attuale provvedimento, l'inserimento dei temi in due o più decreti. In secondo luogo, si potrebbe prevedere l'adozione di forme che possano consentire un ruolo proattivo della Commissione, prevedendo un parere rafforzato, o forme di condivisione e di concertazione dell'*iter* procedurale, quali: audizioni, tempi di presentazione e definizione dei criteri di ammissibilità degli emendamenti con le Commissioni indicate come referenti. Ciò anche per evitare, come è avvenuto, che emendamenti di merito sul provvedimento, presentati dai componenti della Commissione, siano dichiarati discutibilmente inammissibili e quindi, nei fatti, sottratti alla discussione e anche alla riformulazione come possibili ordini del giorno in grado di impegnare opportunamente il Governo. Confido che la sensibilità della Presidenza possa recuperare un'attenzione in questo senso almeno a partire dai prossimi provvedimenti.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, rappresentanti del Governo, il disegno di legge che stiamo esaminando tocca diversi temi importanti alcuni dei quali hanno avuto un notevole impatto sull'opinione pubblica. Ho esaminato, come relatore, questo atto in 10a Commissione collaborando ad esprimere il parere favorevole, per le parti di competenza della Commissione. Sul ripristino del Fondo per lo spettacolo c'è stata una condivisione ampia. Si potrà discutere delle modalità di utilizzo di questi denari, ma la cultura italiana certamente non cammina ancora con le proprie gambe e il sostegno dei privati resta al di sotto dei bisogni. Dunque, bene ha fatto il Governo ad intervenire con urgenza. L'osservazione che, in sede di estensione del parere, ho fatto insieme alla maggioranza della Commissione è stata che sarebbe opportuno cercare forme di finanziamento alternative a quelle previste nel decreto. Credo

dei prezzi a causa della tensioni internazionali che coinvolgono diversi Paesi produttori di petrolio, non sembra un buon segnale per le famiglie collegare il ripristino dei fondi

Aprendo un'altra pagina di questo decreto *omnibus*, desidero esprimere apprezzamento per la speciale attenzione dedicata al più grande scavo archeologico del mondo, quello di Pompei, che è anche una grande risorsa del nostro Paese. Le misure contenute nell'articolo 2, specie il programma di interventi straordinari, sono importanti per ripristinare le condizioni necessarie alla conservazione di questo sito, che è una pagina di storia aperta sotto gli occhi del mondo.

mie competenze), ritengo di particolare importanza l'azione, la volontà espressa dal Governo. La pausa richiesta sarà utile: servirà innanzitutto ad acquisire ulteriori evidenze scientifiche sui parametri di sicurezza degli impianti di produzione di energia nucleare. di produzione di energia nucleare. Si concorda quindi con il Governo sulla necessità di escludere dall'applicazione della moratoria nucleare il parco tecnologico e il deposito nazionale. alla luce dei tragici eventi del Giappone, non possono sfuggire le imprescindibili ragioni di sicurezza che impongono la necessità di avere, nel minor tempo possibile, adeguate infrastrutture al servizio della sicurezza delle popolazioni e dell'ambiente. Senza sicurezza, infatti, si rischierebbe anche un rallentamento del processo di smantellamento delle vecchie centrali tuttora esistenti sul territorio nazionale. Credo anche sia saggio convocare una conferenza nazionale sull'energia, come ha dichiarato recentemente in Aula il ministro Romani, e svolgere l'indagine conoscitiva autorizzata dalla Presidenza del Senato e promossa dalla 10a Commissione, tesa proprio ad ad approfondire il tema della sicurezza degli impianti di produzione nucleare. C'è un punto di questo decreto che è stato preso di mira da una certa parte dell'informazione, il divieto per le società televisive che hanno conseguito ricavi superiori all'8 per cento del valore economico del sistema integrato delle comunicazioni (SIC) di acquisire, prima del 31 dicembre 2012, partecipazioni in imprese editrici di giornali quotidiani. Si è parlato di abito su misura fatto per imbrigliare qualcuno, l'esigenza di tale proroga è stata evidenziata anche dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che ha raccomandato di allineare questi termini al completamento della transizione al digitale terrestre, fissato entro il 2012.

televisione ed elettronica. Ed è giusto che sia così, per non fare un favore a qualcuno, lasciandolo fuori da tale divieto. Ritengo importante poi la norma che proroga al 30 settembre 2011 il termine per stabilire il calendario definitivo per il passaggio al digitale e anticipa il termine dell'assegnazione dei diritti relativi alle frequenze radiotelevisive al 30 giugno 2012. In questa previsione, è opportuno esplicitare il meccanismo per contemperare la ridotta disponibilità di frequenze con il grande numero di operatori locali che le richiedono. Ecco allora l'obbligo per i futuri assegnatari delle frequenze di riservare parte della propria capacità trasmissiva in favore dei soggetti esclusi, facendo sì che nessuna attività commerciale televisiva sia costretta a chiusura. Si sono sollevate critiche sull'articolo 7, che amplia l'operatività della Cassa depositi e prestiti, consentendole l'assunzione di partecipazioni in una vasta gamma di società strategiche per il sistema economico produttivo del Paese e per il sostegno del *made in Italy*, sulla base di un decreto attuativo del Ministero dell'economia e delle finanze. A questo proposito, vorrei rispondere al senatore Agostini, che è della mia Regione, per cui entrambi conosciamo bene quello che succede in Umbria. Egli ha dettato una serie di condizioni; tra queste, mi sembra di aver capito

è una contraddizione interna rispetto alla realtà che conosce il senatore Agostini. Di fatto, è noto a tutti che questo atto serve ad evitare che scalate compiute da operatori esteri possano privare il nostro Paese di attività economiche in settori cruciali dell'economia. Di fronte alla globalizzazione, si deve prendere atto che il capitalismo italiano è ancora debole rispetto a quello statunitense o nordeuropeo, e addirittura a quello cinese, che dispone di capitali ingenti, che va piazzando i propri profitti acquisendo aziende in ogni parte del mondo. Per capire allora il senso di questo articolo 7 bisogna andare forse alla scorsa settimana, all'11 aprile, quando l'assemblea dei soci della Cassa ha stabilito una serie di paletti per eventuali acquisizioni: spicca il divieto - l'ha detto prima il relatore - ad investimenti in società, seppur strategiche, che si trovino in situazioni di crisi economica e finanziaria o rischino di trasferire alla Cassa oneri derivanti da processi di ristrutturazione in corso. Il verbale in cui sono stati enunciati questi principi è stato sottoscritto sia dal Ministero dell'economia, titolare della maggioranza del capitale della Cassa SpA, sia dalle 66 fondazioni bancarie che detengono tutte insieme il 30 Mi pare ci sia poco da dire, o da chiamare in causa oscuri patti di sindacato fra capitalisti, ovvero urlare al neostatalismo o al sindacalismo statolatrico (vero, senatore Morando?).

Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, intervengo in discussione generale sul provvedimento che oggi è all'esame dell'Aula, approvato nei giorni scorsi dal Consiglio dei ministri, chiamato decreto-legge *omnibus*, che agli articoli 1 e 2 prevede il reintegro dei fondi FUS e il sostegno allo spettacolo e ai beni culturali. Ed è proprio con riferimento a questo tema, cioè all'intervento finanziario a favore della cultura, che intendo esprimere alcune considerazioni a nome dell'Italia dei Valori circa l'azione del Governo nazionale e il sostegno della maggioranza. Signor Presidente, siamo ormai da anni in piena emergenza culturale che vede il nostro Paese, giorno dopo giorno, mortificare i tanti lavoratori del mondo dello spettacolo e le tante istituzioni culturali che per noi dell'Italia dei Valori costituiscono un patrimonio imprescindibile. La musica, l'opera, la prosa, il cinema, la danza hanno arricchito questo Paese; le fondazioni lirico-sinfoniche, le orchestre, i cori, le associazioni concertistiche, i teatri stabili di prosa, il grande mondo del cinema, il grande mondo della danza hanno offerto un contributo straordinario a livello culturale ed economico al nostro Paese. Il vostro Governo e l'attuale maggioranza hanno sempre risposto a questo patrimonio con tagli indiscriminati che hanno messo ormai in crisi il sistema. In questi anni, in questi lunghi mesi, accorati sono stati gli appelli di intellettuali, di esponenti delle forze politiche, della società civile, di centinaia di artisti italiani e di lavoratori del mondo dello spettacolo, insieme a tantissimi rappresentanti di istituzioni culturali private e pubbliche, hanno manifestato per far sentire la propria voce e per dire con grande chiarezza che bisognava cambiare rotta. Noi eravamo lì a partecipare alle tante iniziative nei teatri, nelle piazze; contestualmente, eravamo a dire la nostra e a sostenere le loro ragioni nelle Aule parlamentari, per confermare che bisognava cambiare e cambiare in fretta. Proprio nel mese di marzo scorso abbiamo organizzato un convegno a Roma con personalità illustri chiedendo a gran voce l'immediato ripristino dei fondi FUS. Persino il Capo dello Stato più volte ha fatto sentire la sua voce. Oggi, proponete un ripristino parziale (è bene dirlo: soltanto parziale) del Fondo unico per lo spettacolo che certamente non riuscirà a risolvere i problemi che, ormai, con la vostra azione, avete provocato nei confronti delle istituzioni culturali. È, a nostro avviso, imbarazzante che il Governo non sia stato in grado di finanziare questo ripristino con la fiscalità generale, ma abbia dovuto - come si suol dire - mettere le mani nelle tasche dei cittadini con un'imposta di scopo sulla benzina Questo è ormai da anni il vostro modo di operare

È la conferma è il sottofinanziamento dei beni e delle attività culturali, settori che in un Paese civile, come l'Italia, dovrebbero essere ai primi posti nelle voci di spesa. Il tema di fondo resta sempre lo stesso: una sostanziale debolezza delle politiche culturali e una subalternità di queste nei confronti delle politiche economiche e di bilancio.

partire una nuova stagione, in cui le politiche pubbliche devono assumere il tema della cultura come elemento centrale di attenzione per l'azione di un Governo credibile; la nuova stagione deve avere un nuovo passo in cui l'intervento pubblico nel settore della cultura, della musica lirica e sinfonica, della prosa, della danza, del cinema deve essere considerato un vero investimento. *(Applausi

trasferisca a chi di dovere questa protesta, che faccio non in quanto senatore, ma in quanto Presidente della 8a Commissione, che rappresenta maggioranza e minoranza, ferme a denunciare questa situazione assolutamente assurda.

Trovo altresì interessante ed originale quanto disposto dall'articolo 4, che aiuta lo sviluppo tecnologico del nostro Paese, perché con la fissazione di criteri che considerano le dimensioni aziendali, occupazionali e di copertura delle emittenti, si potrà procedere

Credo che tutto questo aiuterà lo sviluppo economico del nostro Paese, perché è a tutti nota l'importanza fondamentale per la nostra finanza pubblica dei ricavi dell'asta delle frequenze, che recenti studi sembrano ipotizzare

Identificati questi criteri, credo saranno premiate. Ma non possiamo neanche dimenticare che offrire a queste imprese le frequenze del digitale non significa zittire o oscurare le altre imprese locali minori, che avranno altre

l'ulteriore misura in grado di garantire la continuità a un comparto fondamentale per la programmazione legata al territorio. In questa norma leggo la coerenza di una scelta che va nella direzione di tutelare

Sono infondati se si ha la pazienza di esaminare l'applicazione che della nuova disposizione del decreto-legge è già stata data con le modifiche dello Statuto approvate all'unanimità

abilita la Cassa ad assumere partecipazioni in società di rilevante interesse nazionale, dunque in possesso dei requisiti a tal fine determinati dall'apposito decreto che dovrà adottare il Ministro Tremonti; ma aggiunge che dovrà trattarsi di società «in stabile situazione di equilibrio finanziario, patrimoniale ed economico» e che «siano caratterizzate da adeguate prospettive di redditività».

e assolutamente rilevanti, sufficienti di per sé ad escludere che la Cassa possa compiere operazioni di salvataggio di imprese decotte o in crisi. Su questo credo che siamo d'accordo. ad escludere l'ipotesi, cavalcata da qualche giornale, che in questo momento il Parlamento sta per varare un fondo "salva imprese" e ogni richiamo all'operatività della GEPI. Vi è però una cosa in più, che forse è sfuggita a coloro che si sono esercitati in questa critica. C'è una dichiarazione congiunta, sottoscritta lo stesso giorno dell'approvazione della riforma statutaria, dall'azionista di maggioranza (il Ministro dell'economia e delle finanze) e dagli azionisti di minoranza (tutte le 66 fondazioni bancarie, che credo non stiano lì a dormire lasciando fare al Ministro ciò che vuole), inserita nel verbale dell'assemblea. Gli azionisti hanno anche voluto ulteriormente precisare, con una sorta di interpretazione autentica, le responsabilità degli amministratori e i criteri da eseguire nelle scelte di investimento che gli organi della Cassa dovranno

in ragione della peculiarità delle nuove forme di intervento introdotte nel rispetto delle finalità istituzionali della Cassa depositi e prestiti».

e in ogni caso avvengano nel rispetto delle disposizioni che presiedono all'esercizio dell'attività della Cassa depositi e prestiti secondo criteri di corretta gestione e redditività». Senatore Agostini, alla fine del suo intervento lei ha citato una cosa che non esiste. Non abbia queste preoccupazioni. In questo decreto-legge, nello Statuto, nessuno ha mai parlato di interventi del fondo, della Cassa, a favore di banche, perché le banche non sono le imprese ricomprese in questo decreto-legge che si vuole esaltare nell'operatività di tenuta... non dice che è possibile fare interventi a favore delle banche. Non lo dice la legge, e lo Statuto è entrato ancora di più nel dettaglio,

della produzione legislativa delle fondazioni bancarie: oggi -ahimè! - tutti i critici di allora sono scomparsi. Tutti sono pronti a sostenere che sono investitori istituzionali seri, che fanno il bene del nostro Paese, ma non si erano accorti, allora, che il regolamento attuativo delle fondazioni

Credo debba essere chiaro a tutti che, da una parte, si esclude in modo incontestabile che l'intervento della Cassa possa servire a salvare aziende in crisi; dall'altra parte, si sottolinea il ruolo dell'intervento della Cassa come strumento di promozione del rafforzamento del nostro sistema produttivo, di sostegno alla capitalizzazione e agli investimenti delle nostre imprese, di supporto alla loro internazionalizzazione. Che cosa avviene nell'operatività indicata dalla legge, dallo Statuto È chiaro che si è voluto distinguere l'impegno e i ruoli della politica, e quindi del Governo, del Parlamento e del MEF, e la responsabilità degli amministratori della Cassa depositi e prestiti. Alla politica spetta determinare il perimetro delle imprese di interesse nazionale, ma non valutare il merito dell'investimento. Agli amministratori della Cassa compete accertare, attraverso opportune *due diligence*, l'effettiva ricorrenza delle condizioni di sostenibilità economico-finanziaria e le adeguate prospettive di redditività dell'investimento. Di ciò gli amministratori risponderanno di fronte agli azionisti, ciascuno dei quali dispone

Governo, colleghi relatori di maggioranza e di minoranza, svolgo questo intervento per segnalare due argomenti di particolare gravità contenuti in un testo chiamato *omnibus*, prassi costante

Vorrei introdurre qualche spunto, e non per spirito di parte, ma per dare un contributo ad evitare qualche disastro. L'articolo 3 L'articolo 3 non è quello che è stato decantato, ossia proroga del divieto di incroci tra stampa e televisione.

Quell'ordine del giorno evocava la necessità di protrarre quel divieto superando la data del 31 dicembre 2012, ossia la proroga di quel termine.

pone la necessità di introdurre nuovi criteri per l'Antitrust, termine generale che io per semplicità evoco affinché si riassuma il tutto. È chiaro che nella stagione multimediale che stiamo vivendo andranno trovati altri meccanismi rispetto alla conta esatta delle reti e delle testate, una conta che fu propria della stagione analogica. Infatti, dopo il 31 dicembre 2012, quando si sarà concluso il passaggio dall'analogico al digitale, dovremo ragionarci che non si commetta qualche forzatura, oltretutto aleatoria o furba, a seconda di come la si valuti.

*antitrust*. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nei giorni passati non è riuscita infatti a stabilire l'ammontare esatto della pubblicità, che di tutte le voci del SIC è quella di più certo calcolo,

abbia qualche ambizione di rigore? Da qui nasce il mio invito a ripensare seriamente questo articolo e di tornare all'ordine del giorno e al suo significato, cioè lo spostamento di un termine puro e semplice ragionando insieme su altre forme normative.

che il Governo si interrogasse seriamente. In uno degli emendamenti presentati noi proponiamo l'abrogazione di questo articolo, nella speranza che si possa discutere di un argomento così delicato. Provo a riassumere

Pioveranno ricorsi, e questo termine si trascinerà all'infinito. Intanto, qui si propone una graduatoria tra le emittenti che ha un unico precedente, che finì alla magistratura tanti anni fa; le graduatorie sono molto insidiose quando non c'è una regolazione precisa e, infatti,

Perché togliere all'emittenza locale dando luogo ad una situazione di restrizione proprio di quei bacini locali che sono nel globale - non per caso si è coniato un valore aggiunto importante, soprattutto nella stagione multimediale? Perché mai rischiare di non fare la gara, ancora una volta, per una scelta di accentuato conflitto di interessi per dare tutto

una cortesia, rivolgo quasi una preghiera, affinché non vengano presi come un semplice dibattito tra Governo, maggioranza e opposizione, perché si gioca una partita molto rilevante per lo stesso futuro del settore.

nel mio intervento vorrei soffermarmi innanzitutto sulle misure di razionalizzazione dello spettro radioelettrico contenute in un lunghissimo, nonché poco chiaro, comma unico dell'articolo 4. Il tema della gestione dello spettro è venuto acquisendo in questi anni un'importanza crescente e, contemporaneamente, è cresciuta la consapevolezza che le frequenze sono in tutto e per tutto assimilabili ad una risorsa naturale. L'elevata richiesta da parte degli operatori e la poca disponibilità della stessa hanno fatto sì che essa divenisse una risorsa scarsa. È nata così l'esigenza di migliorare la gestione delle frequenze. Ricordo che nel 2008, sulla rivista «Quaderni di Telèma», si affermava già che, accanto ai «petro-dollari», si sarebbe parlato sempre più spesso di «radio-euro». Si discute del fatto che il collasso dello spettro radio provocato dall'alluvione di dati mobili è sempre più vicino. Tutto il mondo sta cercando di affrontare l'emergenza, dagli USA all'India. Anche la Commissione europea spinge per prevenire il crollo e stimolare un settore che - come dicevo prima - porterà grandi vantaggi all'economia complessiva. Il commissario all'agenda digitale Kroes ha affermato che entro il 2012 l'uso delle frequenze deve essere armonizzato a livello europeo ed entro il 2013 la banda a 800 megahertz deve essere resa disponibile. È facile capire che a livello internazionale i tempi stringono, ma il problema è che in Italia il Governo ha deciso di accelerare ancora di più. Lo ha fatto con la legge di stabilità e con la necessità di incassare dall'asta (delle frequenze) quei 2,4 miliardi con cui si conta di salvare il bilancio pubblico. Una scelta molto sbagliata, riteniamo noi dell'Italia dei Valori, sulla cui riuscita non sono in molti a scommettere. Recentemente, l'associazione europea degli *other licensed operators* (OLO) - ossia tutti gli operatori di reti di telecomunicazione - ha lanciato un avvertimento sulla questione delle aste, affermando che «i Governi pensano solo a battere cassa», mentre la priorità dovrebbe essere quella di aumentare la concorrenza e quindi avvantaggiare i consumatori. Eccezion fatta per l'Olanda, le aste per il dividendo digitale, nei Paesi in cui si sono già svolte, favoriscono solo i grandi operatori e tendono ad escludere i nuovi entranti. Questo accadrà con la norma che avete deciso di inserire in questo decreto-legge. L'articolo 4 differisce il termine per stabilire il calendario definitivo per la transizione alla trasmissione televisiva digitale terrestre. Inoltre, viene dettata una nuova disciplina di assegnazione delle frequenze radiotelevisive. Voglio ricordare che non sono mancate perplessità anche da parte del Quirinale sulla necessità di inserire in un provvedimento d'urgenza una norma che prevede un meccanismo complesso di graduatorie regionali e, nei fatti, una sorta di esproprio del diritto d'uso delle frequenze nei confronti di una parte dell'emittenza locale. Diciamolo pure, questa è una vera e propria umiliazione delle TV locali, come già detto da altri colleghi. L'obiettivo della norma è, dunque, quello di liberare una banda di frequenze da mettere all'asta. Le frequenze da liberare, i canali dal 61 al 69 della banda UHF, nelle Regioni digitali sono stati tutti assegnati alle emittenti locali e non alle TV nazionali. Sarà stato un caso? Io credo di no. Ci tengo a ricordare che il digitale terrestre era nato proprio per superare la concentrazione esistente e consentire l'emersione di nuovi soggetti e nuovi linguaggi. Stiamo assistendo, invece, purtroppo, alla ripetizione delle stesse logiche che hanno guidato la televisione analogica. Nelle aree dove c'è ancora la TV analogica i canali dal 61 al 69 non saranno quindi più assegnati. Il calendario del passaggio al digitale sarà rivisto entro il settembre 2011. Nelle Regioni digitali, ai soggetti in posizione utile nelle graduatorie regionali saranno dati altri canali nella banda VHF e nella restante banda UHF. Le televisioni nazionali non vengono mai citate nella norma. A saltare sarebbe così la prescrizione di legge che riserva alle TV locali un terzo delle frequenze televisive. L'articolo 4 prevede la formazione di graduatorie per ogni Regione o area tecnica dei soggetti che ne facciano richiesta sulla base di quattro parametri: base di quattro parametri: patrimonio al netto delle perdite; dipendenti a tempo indeterminato; ampiezza della copertura della popolazione; priorità cronologica d'insediamento nell'area regionale. A fronte della condivisione della necessità di liberare frequenze che potranno essere utilizzate per offrire servizi di banda larga *wireless*, desta perplessità proprio la delineazione dei criteri scelti. Infatti se, per esempio, i primi due punti sono senz'altro rappresentativi di una certa dimensione dell'impresa televisiva locale, i due punti successivi potrebbero penalizzare ingiustificatamente alcune imprese che, pur dotate di risorse patrimoniali e di capacità imprenditoriale, operano in aree estese dal punto di vista del territorio, ma a scarsa densità abitativa. Così come il criterio della priorità cronologica rischia di bloccare l'ingresso dei cosiddetti nuovi entranti.

Con la norma al nostro esame si cerca di anticipare i tempi e quindi di arrivare allo *switch-off* nei primi mesi del 2012. A parte la tentazione di bloccare la strada al *competitor* principale di RAI e Mediaset, ossia Sky, che sul digitale ha ancora bisogno di tempo per attrezzarsi, non si può tralasciare che il digitale presenta molti problemi irrisolti nelle Regioni in cui il passaggio c'è già stato. Siamo dunque in una situazione di totale caos. Secondo un articolo pubblicato su «Milano Finanza», si parlerebbe già - prima ancora di convertire il decreto - di uno slittamento breve per lo svolgimento della gara e per il conseguente incasso, anche solo di un paio di mesi rispetto al limite fissato al 30 settembre. È evidente quindi - è la nostra riflessione - che brancoliamo nel buio, che il piano del Governo è fatto solo di iniziative sparse e promesse non mantenute. L'Italia è l'unico Paese europeo a non avere un'agenda digitale condivisa. Manca una cabina di regia. L'unico problema da affrontare per voi è quello della TV. Tutto il resto viene definanziato: stampa, editoria, Internet. Il «Piano Caio» che prevedeva 800 milioni per il superamento del *digital divide* non ha visto un euro. I fatidici 800 milioni sono spariti: a disposizione ce ne sarebbero un centinaio, ma il milleproroghe ne ha già destinati 30 al completamento dello *switch-off*. Questo è il quadro complessivo

nel mio intervento vorrei evidenziare quanto questo provvedimento prevede sulla moratoria sul nucleare. sul nucleare. L'articolo 5 prevede una moratoria di un anno per quanto riguarda le procedure che attengono alla localizzazione e alla realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica nucleare. nello stesso articolo, al comma 2, leggiamo che questa sospensione non si applica per quanto riguarda la localizzazione, la costruzione e l'esercizio del parco tecnologico e del deposito nazionale. È chiaro che la norma, così come è stata strutturata, fa nascere il legittimo sospetto - e anche qualcosa di più - che il Governo che il Governo Berlusconi in realtà non voglia assolutamente dismettere l'idea di una politica nucleare, nonostante la tragedia di Fukushima e

temendo un risultato positivo del *referendum* contro il nucleare promesso dall'Italia dei Valori), sancire una pausa di riflessione; però, è chiaro che, lasciando impregiudicata la parte relativa al parco tecnologico e all'unico deposito di scorie radioattive, faccia pensare che il percorso sarà tutt'altro.

è una questione che in molti Paesi non è stata trattata come penserebbe di farlo il Governo Berlusconi, cioè realizzando un unico deposito di scorie radioattive.

quanto meno, un progetto molto difficile da realizzare nel nostro Paese. Soprattutto, il Governo Berlusconi ha pensato di realizzare un solo deposito senza neanche aver fatto concretamente e in modo approfondito delle indagini sul nostro territorio per sapere se geologicamente ci possiamo permettere di ospitare un deposito come questo. Voglio ricordare che da 30 anni gli Stati Uniti d'America

Con recenti provvedimenti il Governo Berlusconi ha lasciato il compito di localizzare e realizzare il deposito delle scorie, anziché ad un'agenzia pubblica (che,

Potrei trattare altri temi, ma il tempo a mia disposizione sta finendo. Voglio concludere dicendo che mi pare che questa presa di posizione del Governo Berlusconi sia, ancora una volta, una presa in giro degli italiani, che si ritroveranno fra un anno, finita la moratoria, di nuovo con un piano energetico che guarderà solo ed esclusivamente all'energia nucleare. Spero che con il *referendum* che si terrà nel mese di giugno gli italiani possano, ancora una volta, esprimere, come peraltro hanno già fatto diversi anni

il bilancio interno del Senato; ci è stato sempre risposto che era in fase di definizione. La VICE presidente Bonino, la settimana scorsa, ci ha informato che era stato adottato dal Collegio dei senatori Questori e che era il Consiglio di Presidenza a dover

alla fine dell'anno scorso siamo stati informati, senza nessuna consultazione preventiva, che magari avrebbe potuto portare a conclusioni ancora più significative o sensazionali, relativamente alla decurtazione di 1.000 euro

proposta qualunquista, solo che avrebbe dovuto essere inclusa all'interno di un dibattito in cui soppesare gli argomenti a favore e quelli contro. Sicuramente un argomento a favore del contenimento della spesa pubblica ci viene dalla contingenza generale del Paese e anche mondiale; ancor di più ci sarebbe venuto un anelito riformatore, e comunque anche "risparmioso", se avessimo saputo come negli anni - e magari in queste ore - sono stati spesi i soldi interni del nostro Senato. Tutto ciò non è possibile perché siamo arrivati al 18 aprile il documento non è ancora conosciuto. Il documento deve poter essere non soltanto letto ma studiato in maniera approfondita, perché, se non altro, nel piccolo *divertissement* che si verifica quando c'è il dibattito, i documenti che si vengono ad elaborare possano avere un minimo di merito, oltre che fare una serie di denunce demagogiche, come spesso sono quelle che si sentono arrivare dal Gruppo dell'Italia dei Valori. L'anno scorso abbiamo discusso il bilancio preventivo a settembre: sfido qualsiasi consiglio di amministrazione a rinnovare la fiducia ad un amministratore delegato che proponga a settembre il bilancio preventivo. Oggi siamo già a metà aprile e ancora di questo

Il giorno 30 marzo rivolsi al Presidente del Senato una richiesta di intervenire affinché potessimo avere una risposta dal Ministro, perché proprio quel giorno,

questi 1.240 rapporti di lavoro per consentire al Governo di avere il tempo materiale per risolvere con un provvedimento il problema. Questo ha creato in quei 1.240 lavoratori e in tutti noi una grande attesa e speranza.

La esorto, signor Presidente, a chiedere al ministro Sacconi di venire in Aula a riferire su questo fatto, che è grave,